con le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi tre ore, incluse le dichiarazioni di voto.

hanno provveduto a trasmettere alla Presidenza le designazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, per il rinnovo di cui all'articolo 21,

Signor Presidente, onorevoli senatori tutti, oggi in quest'Aula voglio ricordare il tragico incidente ferroviario avvenuto in Puglia quattro anni fa. Alle ore 11 del 12 luglio 2016 si scontrarono due treni lungo la linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Corato e Andria: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite, in uno dei più gravi incidenti avvenuti in Italia, una ferita che resta ancora aperta. Al momento dell'incidente i due treni si trovavano lungo un tratto di ferrovia a binario unico, sul quale non era utilizzato un sistema automatizzato di blocco dei treni. Immagini strazianti che nessuno potrà mai dimenticare, come nessuno potrà mai dimenticare la richiesta di verità e giustizia che proviene dalle famiglie delle vittime cui, come Stato e come istituzioni, abbiamo il dovere di dare risposta, un dovere di chiarezza, di verità e di giustizia che dobbiamo alle vittime, ai loro cari, ma anche a tutti i cittadini italiani. La sicurezza è un tema cui non possiamo e non dobbiamo venir meno. Pertanto, ogni anniversario deve rappresentare un volano, non solo della ricerca della verità, ma anche dell'impegno per la prevenzione, assicurando continui controlli sulle linee ferroviarie. Come diceva sant'Agostino, coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti. Sono degli invisibili e tengono i loro occhi, pieni di gioia, puntati nei nostri, pieni di lacrime. Sono e sarò sempre vicina a tutte le persone che quel giorno furono coinvolte. A loro e a tutti i familiari delle vittime porgo il mio personale sostegno e cordoglio, affinché nessuno dimentichi.

di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ciascun senatore riceverà una scheda di colore giallo, sulla quale indicherà un solo nominativo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione prevista dall'articolo 153, 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Saranno proclamati eletti i due candidati che otterranno il maggior numero di voti. L'elenco delle candidature pervenute, pubblicate nel sito Internet del Senato, è a disposizione degli onorevoli senatori. Per l'elezione di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascun senatore riceverà una scheda di colore rosa, sulla quale indicherà un solo nominativo. Saranno proclamati eletti i due componenti che otterranno il maggior numero di voti. Per le operazioni di voto sono state approntate due cabine dinanzi al banco della Presidenza. I colleghi senatori, chiamati in ordine alfabetico, riceveranno dagli assistenti parlamentari, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, le due schede che, dopo il voto, depositeranno nelle apposite urne all'uscita delle cabine stesse. Ricordo che il risultato non verrà proclamato immediatamente, poiché i senatori che non hanno partecipato al voto potranno transitare sotto il banco della Presidenza e, comunicando il proprio nominativo ai senatori Segretari, deporre le schede nelle urne predisposte. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista per le ore 13,30. Concluse le operazioni di voto, si procederà agli scrutini. Dichiaro aperte le operazioni di voto a scrutinio segreto e invito i senatori Segretari a procedere all'appello.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020». Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Speranza. Signor Presidente, a distanza di un mese dalle mie ultime comunicazioni al Parlamento, sono qui in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, come modificato e approvato dalle Camere. Esso prevede che il Governo si confronti con il Parlamento per informarlo del lavoro svolto e dei suoi orientamenti rispetto ai prossimi provvedimenti. Sono qui per ascoltare con la massima attenzione e preventivamente le valutazioni, le proposte e gli indirizzi che il Parlamento riterrà opportuno proporre all'Esecutivo. Abbiamo iniziato il 4 maggio la fase di uscita dal *lockdown*. Da allora proseguiamo con prudenza il nostro percorso di riapertura. Dentro questo cammino considero rilevante il dibattito parlamentare di oggi. Un confronto è certamente necessario per riflettere sullo stato di evoluzione della pandemia in Italia e nel mondo e per ascoltare le valutazioni e le indicazioni che il Parlamento vorrà esprimere sulle prossime decisioni da adottare. Questa nostra discussione per me non è mai semplicemente un atto dovuto nel rispetto di una norma, ma è una possibilità vera per favorire una corretta dialettica tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione, come ha auspicato autorevolmente più volte il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È con questo spirito che in premessa, prima delle opinioni e delle proposte, voglio partire dalla realtà, dai fatti. Purtroppo, nel corso di questa terribile pandemia abbiamo tragicamente imparato che la realtà e i fatti non sempre coincidono con i nostri desideri e spesso prendono sentieri imprevedibili. Pochi numeri e la loro sequenza sono quasi sempre più chiari ed espliciti di mille parole. Il 31 maggio, quando l'Italia era già nella fase di uscita dal *lockdown*, nel mondo avevamo 5.934.936 contagiati e 367.166 deceduti. Oggi, a distanza di poco più di quaranta giorni, i contagiati hanno superato la soglia dei 13 milioni. Sono dunque più che raddoppiati e i deceduti, oramai, sono tragicamente ben oltre il mezzo milione. Di fronte a questi dati, a questi numeri impietosi, è del tutto evidente che non possiamo abbassare la guardia. Non dividiamoci su questo, vi prego. Anche nella comunità scientifica si dibatte

a partire dal lavaggio frequente delle mani: tre semplici regole ma essenziali, che possono farci gestire questa fase di convivenza col coronavirus. Il dato dei contagiati cresce ovunque: negli Stati Uniti siamo oltre i tre milioni e dalle Americhe ogni giorno ci giungono, da più parti, strazianti immagini di dolore e disperazione. L'onda diventa sempre più alta anche nei Paesi orientali e nel sud del pianeta, dove i dati, con un sistema sanitario molto fragile, sono purtroppo spesso incompleti e parziali, dentro un vortice drammatico di numeri e percentuali

nel nostro pianeta, ad oggi, il Covid ha colpito un cittadino ogni circa 650 abitanti dei quasi otto miliardi di donne e uomini che popolano la terra sulla quale viviamo. Questa è la straripante forza di un nemico che non solo non abbiamo ancora sconfitto, ma che continua espandersi, occupare altri territori, a mietere nuove vittime; un virus subdolo, che spesso colpisce mimetizzandosi. il Covid ci attacca moltiplicando i contagiati non solo attraverso soggetti sintomatici, ma sempre di più per mezzo di pazienti Ricordo questi numeri non per alimentare paure irrazionali che non avrebbero alcun senso, ma per non smarrire la razionale consapevolezza

Conosciamo sempre di più il virus e abbiamo adottato misure di prevenzione territoriale, nei luoghi di lavoro, come protocolli di sicurezza negli ospedali e nelle nostre strutture sanitarie. Non facciamoci illusioni, però: non esiste il rischio zero senza il vaccino. Io credo che tutto il Parlamento, tutti gli italiani debbano essere consapevoli del lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di mettere alle spalle i giorni più bui. Come ho già detto in precedenti interventi in quest'Aula, dobbiamo riconoscerlo e valorizzarlo, come fa, d'altronde, larga parte della comunità internazionale, ma senza chiudere gli occhi dinanzi a quello che non ha funzionato, come sarebbe stato necessario. Non ci ha regalato niente nessuno. Per primi, in Occidente, siamo stati Ci siamo misurati con difficoltà e problemi inediti per tipologia e dimensioni. Abbiamo combattuto con coraggio e determinazione, senza avere un manuale d'istruzione da consultare per orientare le nostre scelte. Quale fosse la scelta giusta, in ogni singolo passaggio, non c'era scritto da nessuna parte. Quando uso il plurale, il mio non è un plurale riferito al Governo Mi riferisco all'Italia, alla nostra Nazione nel suo insieme. Mi riferisco a tutte le istituzioni repubblicane: Governo, Regioni, Comuni, Province e soprattutto agli italiani, che hanno svolto un ruolo determinante, facendo sacrifici inimmaginabili; al personale sanitario, alle forze di polizia, ai volontari e ai lavoratori che, per assicurare i servizi essenziali, hanno continuato a svolgere le proprie attività anche durante il *lockdown*. Non finiremo mai, mai, di ringraziare quelle donne e quegli uomini.

Abbiamo indicato una rotta di navigazione nella tempesta, che poi è servita ad altri ed è seguita oggi da quasi tutto il mondo. Lo dico con grande dolore nel cuore. Chi ha fatto scelte differenti dalle nostre, chi si è affidato all'ipotesi dell'immunità di gregge sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane ed è ancora pienamente dentro la tempesta. Noi, l'Italia, oggi siamo fuori dai giorni più drammatici della tempesta. Viviamo in un mare poco mosso, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Non siamo ancora al riparo, per due motivi, tanto semplici quanto evidenti. Il primo il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. Siamo dentro una fase di convivenza con il Covid, in un contesto nel quale, aumentando le attività e liberalizzando gli spostamenti, aumentano, inevitabilmente, le probabilità di incontrare il virus. Lo testimoniano i numerosi focolai attivi, che dobbiamo essere sempre più rapidi a individuare e isolare con il massimo della determinazione e senza alcuna alcuna incertezza. Il secondo motivo è che siamo oggettivamente esposti al rischio di importare il virus da italiani che tornano da viaggi all'estero o da cittadini di altri Paesi che arrivano o transitano in Italia. Sono rischi non teorici, ma concreti, che, muovendoci con grande prudenza, possiamo ridurre sensibilmente, ma mai azzerare del tutto. Sono rischi che le nostre rilevazioni settimanali mettono chiaramente in evidenza, pur dentro un quadro nazionale che, anche questa settimana, rileva un indice RT inferiore ad 1.

piccole catene di contagio di cui non sempre è facile riscontrare l'origine. Sia dai dati internazionali che da quelli nazionali, risulta, dunque, confermata la valutazione che la partita per arginare, prima, e sconfiggere, dopo, il Covid è tutt'altro che terminata. Ecco perché dobbiamo muoverci in ogni circostanza ispirati dal principio di massima precauzione, non sottovalutando alcun segnale di pericolo e sempre pronti a intervenire in modo tempestivo e proporzionale all'evoluzione della situazione epidemiologica. Discuteremo nuovamente - sia alla Camera che al Senato - con uno specifico ordine del giorno dell'eventuale proroga dello stato di emergenza. Voglio essere molto chiaro: al momento nessuna decisione è stata assunta. Dovrà riunirsi il Consiglio dei ministri e personalmente sono profondamente che il Parlamento debba essere pienamente protagonista del percorso decisionale nel rapporto di fiducia che lo lega al Governo. Lo stesso Presidente del Consiglio mi ha ribadito la sua piena disponibilità a un ulteriore momento di confronto *ad hoc* sul tema con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati. Con la stessa franchezza, alla luce del quadro che ho precedentemente lineato, credo risulti evidente a tutti che io non considero terminata e archiviata la fase di emergenza. Il punto aperto è discutere di quali siano gli strumenti formali più adeguati per affrontarla. Valuteremo con trasparenza - anche con il confronto con le Camere tutte le ipotesi in campo; nessuna al momento può essere esclusa in termini sia di procedure e conseguenze giuridico-amministrative sia di temporalità. convinto che lo stato di emergenza non possa che essere legato a un periodo eccezionale e limitato della vita del nostro Paese. Quello che ci preme è essere pronti, non avere intoppi o ritardi, poter essere tempestivi nelle procedure, come - ad esempio - le gare per i banchi o per i test sierologici in vista della riapertura delle scuole. Quello che non possiamo permetterci è non avere una macchina efficace e veloce per rispondere a ogni evenienza, perché il rischio c'è e non si può far finta di non vederlo. Credo - permettetemelo - che il tema del rapporto tra epidemia e democrazia meriti un ulteriore momento di approfondimento, anche in vista delle scelte che a breve saremo chiamati a compiere. Dinanzi alle immagini del primo impatto del Covid in Cina, alcuni osservatori hanno immaginato e anche scritto che le regole della democrazia potessero rappresentare un limite per affrontare l'epidemia e fermare il contagio e che invece i Paesi con un forte dirigismo centrale fossero naturalmente più attrezzati per affrontare l'emergenza. Penso che non sia così. Nella nostra esperienza italiana la chiave più importante per piegare la curva del contagio è stata proprio la sintonia di fondo tra le misure che abbiamo adottato e il sentire comune della popolazione, consapevole dei rischi che tutto il Paese stava correndo. non è mai stata la chiave securitaria quella decisiva, ma lo sono state la persuasione e la convinzione delle persone. Penso che la democrazia e le sue regole rappresentino sempre un punto di forza, mai un punto di debolezza, e credo che queste riflessioni valgano anche per i prossimi mesi. In una fase in cui nel mondo viaggiamo al ritmo di oltre 200.000 nuovi contagi al giorno è difficile non riconoscere con linearità e trasparenza che la sfida è ancora aperta per ciascun Paese, nessuno escluso. L'ho ripetuto mille volte in questi mesi e non mi stancherò mai di ripeterlo: il virus non conosce confini regionali, nazionali e internazionali. Sono mille le strade attraverso le quali il contagio può essere importato in Italia e innescare nuovi focolai di infezione. In questo quadro il nostro obiettivo sarà garantire un giusto e proficuo equilibrio tra le preziose e incomprimibili prerogative del Parlamento e l'urgente necessità di tutelare la salute pubblica. Il Parlamento ha definito, con la conversione del decreto-legge n. 19 del 25 marzo, e poi con il decreto n. 33 del 16 maggio, un percorso, una modalità di funzionamento alla quale il Governo - come sta già puntualmente facendo - intende scrupolosamente attenersi. I commi 1 e 5 dell'articolo 2 decreto-legge n. 19 definiscono con chiarezza il procedimento da seguire nell'adozione di misure di contenimento. Dentro questo sentiero la mia opinione è che sia pienamente possibile contemperare e mantenere in giusto equilibrio il diritto fondamentale alla salute, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, e le prerogative che sempre la nostra Carta costituzionale attribuisce al Parlamento. È chiaro che l'Italia è in una fase diversa rispetto ai mesi passati: dal 4 maggio abbiamo cominciato a riaprire e a ripartire con giudizio, ma dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo farlo anche per non pagare un prezzo troppo alto sui piani economico e sociale, ma ai nostri concittadini dobbiamo sempre dire una verità, una verità decisiva e importante. La prima misura, quella più forte per riavviare la nostra economia, è continuare a rispettare rigorosamente tutte le regole di prevenzione adottate, a partire da quelle relative ai nostri comportamenti individuali. Senza la sicurezza sanitaria non ci sono legge di bilancio, investimento pubblico-privato o finanziamento europeo in grado di farci recuperare il terreno perso in questi mesi. Per convivere con il virus sino al vaccino, per riaccendere tutti i motori della nostra economia e per affrontare i gravi problemi sociali che vediamo crescere nel nostro Paese non dobbiamo arretrare di un millimetro sulle misure di prevenzione.

Le principali misure sono: l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi; l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; il divieto di assembramenti; le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena; il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra-UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine. Quest'ultima misura, che ho adottato con mia ordinanza, è direttamente correlata alla grave situazione di contagio in un numero crescente di aree del mondo. La scelta è chiara: non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi ed è per questo che abbiamo scelto ancora una volta la linea della massima prudenza. Il divieto di ingresso e transito in Italia riguarda a oggi chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato e transitato in tredici Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana; sono le Nazioni che hanno un'alta percentuale di incidenza del virus in rapporto alla popolazione e una resilienza molto bassa dei sistemi di prevenzione e di controllo. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell'ordinanza. Aggiorneremo costantemente questa lista sulla base di un'analisi puntuale dell'evoluzione dei dati epidemiologici. che, per tutti gli arrivi dai Paesi extraeuropei ed extra-Schengen, abbiamo confermato la quarantena di quattordici giorni come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Particolare attenzione è rivolta in queste ore agli sbarchi sulle nostre coste, con rigorosi controlli sanitari e obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano. Nessuna sottovalutazione può essere ammessa. Sull'urgente necessità di coordinare e controllare con misure comuni le frontiere europee, nei giorni scorsi ho scritto una lettera al commissario europeo alla salute e alla sicurezza alimentare Stella Kyriakides e al ministro della salute tedesco, presidente di turno, Jens Spahn. Nella lettera ho insistito sull'inderogabile esigenza di definire nuove, rigorose misure cautelative per gli arrivi da aree extra-Schengen ed extra-UE, richiedendo a Commissione e Presidenza di promuovere un maggior coordinamento tra gli Stati membri e garantire così una maggiore efficacia alla realizzazione dell'obiettivo di contenere la diffusione di contagi causati da focolai di origine esterna. Ogni misura di divieto di ingresso in Italia e di limitazione della libera circolazione dei voli è una decisione che assumiamo con dolore, ma sono scelte necessarie. L'Italia vuole isolare il virus, fermare la catena del contagio e non isolare i Paesi colpiti, nei confronti dei quali riconfermiamo la nostra massima disponibilità di aiuto e di cooperazione. Siamo al lavoro con il ministro degli esteri Di Maio e con il commissario Arcuri per corrispondere positivamente, a partire dal Brasile, alle tante richieste di aiuto che ci giungono da Nazioni particolarmente in difficoltà a causa della pandemia. L'Italia farà fino in fondo la sua parte, nessuno si salva da solo. Un virus globale si batte anche e soprattutto con una forte cooperazione internazionale. *(Applausi)*. Parallelamente a questi provvedimenti, sempre relativamente alla gestione dell'emergenza, il Governo è impegnato tutti i giorni su quattro fronti prioritari, il primo dei Il nostro Paese, l'Italia, è pienamente in campo per assicurare al più presto il vaccino a tutti i cittadini; un vaccino che - lo ribadisco con forza - è per l'Italia un diritto di tutti, un bene pubblico globale, non un privilegio di pochi. Rispetto alla mia precedente informativa, devo sottolineare che l'iniziativa che abbiamo intrapreso come gruppo di testa, insieme a Germania, Francia e Olanda, ha provocato un'accelerazione delle iniziative della Commissione europea su questa partita decisiva per sconfiggere definitivamente il Covid. L'accordo che abbiamo firmato con AstraZeneca prevede la produzione di 400 milioni di dosi, di cui 60 milioni da consegnare entro la fine dell'anno. È una bella notizia che il vettore virale del vaccino di AstraZeneca, su cui ha lavorato *in primis* l'università di Oxford, è fatto a Pomezia e che l'infialamento avverrà ad Anagni: sono segnali che l'Italia c'è. L'Italia c'è, con i suoi cervelli e con le sue competenze. Continua, poi, in questi giorni il confronto con gli altri Paesi europei per chiudere accordi con altri candidati vaccini credibili; interloquiamo a trecentosessanta gradi con tutti i potenziali produttori. Nei giorni scorsi ho visitato prima l'IRBM di Pomezia, poi ReiThera di Castel Romano, dove pure si lavora a un vaccino tutto italiano, e poi, ancora, lo stabilimento Catalent di Anagni, dove anche la Johnson&Johnson, oltre ad AstraZeneca, infialerà il vaccino in sperimentazione. *(Applausi)*. L'Italia ha enormi potenzialità connesse all'industria farmaceutica e questo è un *asset* strategico del Paese. Dobbiamo valorizzare i siti italiani in grado di produrre e attrarre nuovi investimenti internazionali. È questa la scelta di fondo a cui stiamo lavorando. fronte riguarda gli ospedali Covid. Mi fa molto piacere informare il Parlamento che, entro pochi giorni, entro la fine della prossima settimana, il Ministero della salute avrà terminato l'esame di tutti i progetti pervenuti dalle Regioni per gli ospedali Covid, ai sensi del decreto rilancio; conseguentemente saranno trasmessi al commissario straordinario per l'emergenza, per mettere in essere, con procedure straordinarie, tutti gli adempimenti necessari per la loro più rapida realizzazione. Si tratta di un passo in avanti fondamentale per rafforzare la nostra rete dell'emergenza, delle terapie intensive e sub-intensive e, contemporaneamente, rendere più sicuri i nostri ospedali, superando qualsiasi forma di promiscuità tra la rete Covid e quelle non Covid. all'aumento del personale sanitario e al rafforzamento del territorio. Si tratta di un lavoro senza precedenti: abbiamo investito più risorse sul Servizio sanitario nazionale negli ultimi cinque mesi che negli ultimi cinque anni;

Il prossimo passo, con l'adozione definitiva del decreto rilancio, sarà l'assunzione a tempo indeterminato di 9.600 infermieri di comunità: una svolta storica che ci consentirà di rafforzare concretamente i servizi territoriali, che rappresentano - come anche questa emergenza ci ha confermato - il baluardo fondamentale per prevenire e successivamente gestire le emergenze sanitarie. È particolarmente strategico l'investimento sui servizi domiciliari alle persone fragili, che farà passare l'Italia dal 4 per cento della platea di assistiti *over* 65, al 6,7 per cento; passiamo, grazie a un solo decreto-legge, dall'essere due punti sotto la media dei Paesi OCSE a 0,7 punti sopra la stessa media. L'investimento sul personale è fondamentale sempre e lo è in modo particolare in queste settimane, in cui la nostra priorità deve essere recuperare le visite e gli interventi che sono stati sospesi a causa del Covid. Il coronavirus - come è ovvio non ha fermato le altre patologie, a partire da quelle croniche o ad esempio oncologiche, e ora più che mai il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di più energie per recuperare il ritardo accumulato. Dobbiamo sostanzialmente

Senza la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado non saremo mai completamente fuori dal *lockdown*. Con l'accordo raggiunto il 26 giugno scorso in Conferenza unificata tra Regioni, Province e Comuni abbiamo compiuto un importante passo in avanti, condividendo le linee guida e gli obiettivi da perseguire. È un appuntamento che va gestito con la massima cautela e prudenza, anche alla luce delle tante difficoltà in cui si sono imbattute le Nazioni che prima di noi hanno deciso di aprire le scuole. La riapertura delle scuole riguarderà circa 10 milioni di persone. Tutte le simulazioni fatte a fine aprile per decidere le modalità attraverso le quali procedere a un graduale superamento del *lockdown* indicano nella scuola una delle attività a maggior rischio proprio per l'elevato numero di persone coinvolte. Per questo motivo, dobbiamo concentrare ogni attenzione sulle riaperture di settembre e tenere un livello di monitoraggio su quanto avverrà nei mesi successivi nelle scuole. anzitutto lavorando alla definizione di una strategia organica di prevenzione. Il personale scolastico sarà sottoposto a indagine sierologica il commissario Arcuri ha già bandito la gara per i *kit* - ed è poi allo studio un modello di *test* molecolare a campione per tenere sotto controllo la popolazione studentesca durante il corso dell'anno. La chiave del nostro lavoro è è ristabilire un contatto più stretto tra scuola e dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territoriale. Negli anni dei tagli, con una decisione a mio avviso sbagliata, è stata archiviata la medicina scolastica, che era stata normata nel lontano 1961. I presidi, i professori e il personale scolastico, non possono essere lasciati soli nella gestione di questo difficile passaggio. Per questo è - a mio avviso ricostruire un rapporto strutturato e non saltuario tra scuola e sanità, che purtroppo manca da troppo tempo nel nostro Paese. Il comitato tecnico-scientifico farà a settembre un'ulteriore verifica sulla modalità di ripresa in piena sicurezza delle lezioni, anche relativamente all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento, ovviamente sulla base dell'andamento del contagio. Una cosa a me sembra certa e indiscutibile: le scuole frequentate dai nostri figli e nipoti riapriranno; sono un valore fondamentale del Paese a cui dedicheremo ogni energia e ulteriori ingenti investimenti economici e finanziari. A scuola dovranno esserci misure di precauzione all'altezza della situazione; a scuola si deve poter andare in piena sicurezza. È con questo spirito che intendiamo affrontare le prossime settimane e la ripresa successiva al mese di agosto. Credo che dobbiamo farlo non smarrendo il filo di uno sforzo unitario. So che non è semplice, ma dobbiamo provarci. La ricerca della massima convergenza nella gestione di questa difficile emergenza sanitaria non è una concessione che il Governo regala alle opposizioni, né uno sconto che le minoranze fanno all'attuale maggioranza parlamentare. Per me è semplicemente la via maestra per portare il Paese definitivamente fuori dalla tempesta; è la via della responsabilità, l'unica - a mio avviso seriamente percorribile nell'interesse prioritario e prevalente del nostro Paese. Spero che il dibattito di oggi saprà essere all'altezza di questa sfida.

a tratti addirittura così esaustivo da dare l'idea che forse il difetto principale che si può far rilevare è quella patologia che noi chiamiamo la "completite", cioè voler toccare tutti i punti e voler lanciare un messaggio preciso, puntuale, articolato e io mi auguro verificabile su ognuno dei punti. Questo è quello che talvolta, che talvolta, perlomeno dal fronte dell'opposizione, ravvisiamo come elemento di maggiore debolezza di un Governo che annuncia molte cose, tutto sommato interviene anche per correggere le cose che ha annunciato e in qualche modo gioca sempre un'immagine di sé che vuole essere al *top* delle esigenze. La prima delle osservazioni che mi sento di farle farle è quella relativa al tempo dell'emergenza. Lei oggi è qui con noi per parlare proprio di emergenza e a tale proposito la prima domanda che tutti si pongono è: fino a quando durerà questa emergenza? Lei ci ha già detto giustamente che non si sa, che una decisione ancora non è stata presa, che è una decisione che si prenderà con il Parlamento, ma non le nascondo che tutti noi abbiamo già sentito che l'emergenza durerà fino al 31 dicembre o fino al 30 di agosto; adesso lei ci dice che per ora l'emergenza durerà fino al 30 luglio.

cosa invece ancora non è stato deciso e - lo dico soprattutto per quanto riguarda l'opposizione - quali sono i margini reali per intervenire con un contributo positivo. Lei sa meglio di me, perché arriverà domani in Aula il decreto rilancio, la sofferenza profonda del Senato è quella di essersi sentito radicalmente escluso dal dibattito. Questo glielo diremo domani tante volte, in tanti modi, in tante circostanze, e io ho avuto modo di dirlo oggi in Commissione, ma il Senato sul decreto rilancio non ha potuto "toccare palla",

Ministro, lei più di noi sa quante contraddizioni fino ad oggi hanno accompagnato questo tema. I genitori non sanno cosa accadrà dei propri figli. Il Ministro ha già detto che il 15 per cento dei ragazzi non avrà posto nelle scuole; le madri che hanno inteso iscrivere i bambini piccoli all'asilo statale o comunale si sono sentite dire che non c'era posto per i piccoli di tre anni, si sono avvicinate allora alla

nulla, come pure sulla vita che toccherà ai ragazzi portatori di disabilità, che in questi mesi sono stati totalmente esclusi dalle iniziative della didattica a distanza.

ma i centri di riabilitazione per i ragazzi non sono stati aperti, quindi abbiamo una fascia di gente supervulnerabile che non è stata nelle RSA né è morta di Covid, ma che oggi troviamo molto più fragile e debole di quanto non l'abbiamo lasciata sei mesi fa. Ci sono tante cose belle in quello che ha detto, ma vogliamo fatti,

dalle misure di qualunque tipo, ma i familiari - i famosi *caregiver* - che hanno speso la loro vita in questi sei mesi facendo gli insegnanti, la riabilitazione, i logopedisti, i fisioterapisti e i terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva non hanno avuto nulla. Questa è una fascia di persone, Ministro, che noi le affidiamo specificamente. Concludo, signor Presidente, perché potrei andare avanti ancora molto a lungo: dateci fatti e saremo con voi.

non possiamo più permetterci di essere impreparati qualora

se il Governo, insieme alle Regioni e agli enti locali, abbia di fatto preparato e predisposto un piano di prevenzione pandemica.

ha un piano di prevenzione e, soprattutto, che apre un confronto su questo piano con il Parlamento e con tutti i cittadini rendendolo noto, in modo tale che ognuno sappia come ci si deve comportare di fronte, ad esempio, all'esplosione di nuovi focolai. Possiamo garantire al Paese che non ci sarà un nuovo *lockdown* e che, per contrastare eventuali nuovi focolai verranno, ad esempio, istituite le microzone rosse, perché non possiamo più permetterci di chiudere tutte le imprese? Questo sta scritto da qualche parte? Altra questione. Abbiamo questa volta tutti gli strumenti per garantire protezione ai nostri cittadini? Faccio un esempio: abbiamo fatto scorte di farmaci,

con qualcuno della minoranza che è intervenuto per dire: anziché accusarci gli uni con gli altri - il nostro intervento è prevalentemente costruttivo - cerchiamo di imparare dagli errori che sono stati fatti. Anziché mettere in contrapposizione il Governo con le Regioni all'inizio dell'intervento, per fare in modo che ci sia una sinergia e una collaborazione tra tutti gli enti preposti? Perché se dobbiamo affrontare una pandemia sarebbe stupido mettersi a litigare tra vari enti; lavoriamo tutti insieme a prescindere dall'articolo

facciamo un servizio al Paese. Stiamo facendo questo lavoro coinvolgendo la Conferenza Stato-Regioni e gli enti locali per far sì che questa volta tutti siano in grado di essere preparati ad affrontare la situazione, evitando *lockdown* e problematiche a tutta la nostra economia? tutta la nostra economia? Abbiamo pronta una campagna educativa-informativa che aiuti i cittadini a capire come ci si deve comportare, che non bisogna abbassare la guardia, dove va indossata la mascherina, dove magari si può essere un po' più tolleranti e non metterla? Tutto questo è predisposto in un piano? Queste sono le domande che stiamo facendo. La cosa migliore, per noi che siamo all'opposizione in termini prevalentemente costruttivi, è che il ministro Speranza risponda a questa interrogazione, venga in Aula

allo stato di emergenza. Il 31 gennaio era stato dichiarato lo stato d'emergenza, ma non è che dichiarandolo siamo sicuri di garantire la salute dei cittadini (abbiamo infatti visto quello che poi è accaduto). Non è formalizzando un atto che siamo certi che le cose andranno bene. Qui ci vuole davvero un piano di prevenzione;

La trovo convincente per le ragioni di merito che riguardano la decisione che siamo chiamati a prendere quest'oggi, votando le proposte - lo ricordo a me stesso e ai colleghi - della decisione di prorogare fino al 31 luglio alcune elementari misure di precauzione e regole di base, che si sono rivelate preziosissime fino ad oggi e che io credo debbano rimanere in campo a tutela della salute dei Trovo particolarmente convincente il richiamo che il Ministro ha fatto alla notevole entità dei nuovi contagi giornalieri che ci sono a livello mondiale: 500.000 sono un numero impressionante. Prendere delle precauzioni per quanto riguarda gli arrivi dall'estero non è isolazionismo, ma è una questione di realismo e di opportunità. Credo che queste misure in primo luogo debbano essere prorogate e che sia comprensibile che si proceda in questa direzione. Lo stesso dicasi per le regole di base sull'indossare le mascherine, sulla distanza di di sicurezza, sui divieti di assembramento, sull'importanza che nei luoghi di lavoro si rispettino le norme di sicurezza. Penso che noi dobbiamo avere la consapevolezza di quanto sia importante

Ma, al di là di questo, trovo convincente l'impostazione generale dell'intervento del Ministro, che ci ha ricordato come la nostra linea di prudenza ragionata e ferma e di massima allerta in tutte le fasi dell'emergenza ci ha consentito di rispondere con i fatti a chi ha rivolto critiche poco fondate all'azione del nostro Governo. Nel corso delle settimane, man mano che l'emergenza si evolveva,

credo che non ci sia da preoccuparsi della polemica, a mio avviso poco fondata, di chi sparge accuse di mancato rispetto della Costituzione, di misconoscimento delle prerogative del Parlamento, di volontà di scavalcare le prerogative e le attribuzioni di organi fondamentali dello Stato e di minare l'equilibrio dei poteri. Mi pare davvero una polemica fuori luogo e fuori misura. Le parole del Ministro sono state estremamente rassicuranti ed estremamente chiare e io credo che possiamo affrontare questa seconda fase dell'emergenza, che è senz'altro una fase di rischi meno acuti, pensando che non è finito il tunnel, ma che sicuramente la fine del tunnel pare essere più vicina. vicina. Penso che nella gestione delle misure che debbono essere prese per evitare rischi si possa adottare un principio di proporzionalità e riconoscere che, in circostanze diverse, i margini per un coinvolgimento in primo luogo preventivo, ma anche successivo e di valutazione a consuntivo del Parlamento sono più ampi di quelli che c'erano fino a poche settimane fa. Accolgo quindi con estremo favore l'impegno del Ministro a far sì che

Siamo in una fase contrassegnata da grossi interrogativi e da grosse incertezze. Speriamo di aver imboccato una strada che ci porti rapidamente fuori dal pericolo, ma non possiamo dirci sicuri di questo. In una situazione del genere non si deve fare niente di più di quello che è necessario in termini di prevenzione, ma nemmeno niente di meno. Credo che il Governo debba tenere questa linea, nel pieno rispetto del Parlamento e mantenendo l'impegno a un'informazione preventiva quando si dovranno approvare degli atti importanti. importanti. Ritengo anche convincente il fatto che sia in corso una valutazione sul tipo di strumento più appropriato da adottare per fronteggiare i nuovi rischi che abbiamo davanti. Non dividiamoci in fazioni e in dispute ideologiche che oggi riguardano lo stato di emergenza e domani un'altra cosa: cerchiamo di ragionare per obiettivi; fissiamo l'obiettivo, definiamo la necessità e poi scegliamo tutti insieme, senza escludere nessuno e senza violentare le prerogative di nessuno, lo strumento più appropriato. Credo che se seguiamo questa linea potremo continuare a ottenere risultati importanti. Ovviamente, anche in questo caso, è necessario sottolineare che per l'ottenimento dei risultati il senso di responsabilità dei cittadini e la grandissima passione e dedizione al lavoro di decine di decine di migliaia di operatori sanitari sono stati fondamentali, insieme alla lucidità di chi ha dovuto prendere le decisioni più delicate.

È vero dunque che la battaglia non è vinta e il virus continua a circolare, ma in considerazione del fatto che i virologi di cui si fida sostengono che il virus sarà sconfitto solo quando avremo il vaccino, mi chiedo se è intenzione sua e del Governo prorogare le misure che ci ha appena elencato fino a quando non arriveremo a tale soluzione: saremmo l'unico Paese al mondo. Sa bene quanto per Forza Italia sia importante la tutela della salute dei cittadini e degli operatori sanitari, che non smetteremo mai di ringraziare e che ancora oggi sono in prima linea negli ospedali; conosce altresì la nostra disponibilità alla collaborazione, ma da politico a 360 gradi non crede ci si debba fidare un po' di più degli italiani e molto meno di chi in questi mesi ha rocambolescamente cambiato idea troppe volte? Consiglio dei ministri appena illustrato ci sarebbe stata la possibilità di aprire, di allargare, perché se continuiamo a restare chiusi le nostre città muoiono, i cittadini soffrono la mancanza di lavoro e la libertà di poter percorrere le nostre strade senza dover pensare di essere sempre penalizzati per colpa dell'incuranza di altri. Ci saremmo aspettati che si fidasse un po' più del politico che è in lei piuttosto che, ancora una volta, del comitato tecnico-scientifico,

Ci saremmo aspettati che lei potesse decidere, naturalmente con coscienza e seguendo i tecnici, ma pensando anche a come comportarsi per il bene del Paese. È vero, i messaggi che arrivano dal Governo fanno pensare, soprattutto negli altri Paesi europei, che l'Italia continui a essere a rischio, perché noi sappiamo anche che la risalita dell'indice di contagio è dovuta in primo luogo a una mancanza di controllo anche dei migranti che arrivano dalla rotta dei Balcani: sappiamo che in Emilia-Romagna e nel Lazio sono aumentati per tutti i contagi dei lavoratori rientrati dal Bangladesh. La politica del massimo rigore l'abbiamo apprezzata certamente quando i nostri ospedali erano stracolmi di pazienti in terapia intensiva, ma forse adesso è il caso di applicare quel massimo rigore per la tutela della salute ai confini delle nostre coste. Quali protocolli, quali controlli sono previsti per queste navi in arrivo? Cosa pensa dell'allarme lanciato dai servizi segreti italiani sul possibile sbarco sul nostro territorio di almeno 20.000 immigrati provenienti dalla Libia? Continuate a permettere alle organizzazioni non governative di farli sbarcare e agli scafisti di guadagnarci? Abbiamo le strutture idonee a contenere il contagio con la popolazione residente o dobbiamo aspettarci che nelle Regioni del Sud, che per fortuna non hanno avuto picchi altissimi di pazienti Covid, si riempiano gli ospedali e le terapie intensive? Quell'errore fatto all'inizio, quando si diceva che sarebbe andato tutto bene, che il nostro Paese era prontissimo e non occorreva avere alcuna paura, lo dobbiamo ripetere per forza o è il caso di predisporre un piano che tenga conto di possibili situazioni sanitarie emergenziali con l'arrivo di ulteriori clandestini? Penso che sarebbe il caso di presentare un piano pandemico. Il primo piano pandemico è stato presentato dal Governo Berlusconi nel 2005 per l'aviaria, aggiornato nel 2009 per l'influenza suina, poi il buio: non c'è ancora, eppure è da gennaio-febbraio che siamo in questo stato e un piano per la pandemia questo Governo non l'ha ancora aggiornato, né soprattutto presentato! Ora, visto che non è possibile predisporre un piano o almeno piccole cose per l'arrivo dei clandestini, si dia ai presidenti di Regione la possibilità di decidere se autorizzare le feste di paese o l'apertura delle discoteche, ma dia loro anche la possibilità di tutelare i propri cittadini e quelli che ancora vorrebbero, magari, andare in vacanza con le famiglie senza rischiare di prendere la Covid perché i centri di accoglienza sono fuori controllo. Non mi permetterò di commentare quanto i giornali hanno scritto rispetto all'ipotesi di decidere di far slittare alla fine dell'anno lo stato di emergenza, legittimando restrizioni personali alle quali noi siamo decisamente contrari. Comunque ci sarà modo e maniera per farlo con il presidente Conte che speriamo venga in Aula a spiegare chiaramente le ragioni che spingono a questa scelta importante. Quello che vorrei da lei, Ministro, è un atto di coraggio. Lo stesso che ha fatto per chiudere gli ingressi a chi proviene dai Paesi più colpiti e che hanno fatto nascere nuovi focolai nel nostro Paese.

Le nostre proposte, anche sul piano della sanità, gliele abbiamo illustrate più volte. L'acronimo MES, tanto odiato da una parte della maggioranza, potrebbe essere utile anche in tal senso. La prego, non si faccia contagiare dal virus della demagogia e del populismo, ma si faccia portatore degli stessi valori del nostro servizio sanitario per la tutela della salute dei cittadini che vogliono continuare a vivere in un Paese libero e democratico. *(Applausi)*.

e quando ci sarà la proroga dello stato di emergenza, se e quando coinvolgerete il Parlamento e in che modalità. Non ho sinceramente neanche capito quali siano le motivazioni e le ragioni tecnico-scientifiche sulle quali poi baserete le vostre decisioni. Chi vi fa da consulente, i membri licenziati che appartengono alle *task force* ai comitati? Quelli che suggeriscono l'utilizzo di *app* che poi vanno a monitorare gli stili di vita, i consumi e lo stato di salute, in attesa di un vaccino che non si sa se mai ci sarà? Infatti il virus ha avuto, secondo gli ultimi studi dell'Imperial college, circa 200 mutazioni. Oppure fate riferimento e avete a supporto quegli scienziati che dicono che il virus è nell'aria? Ma in tutto questo, Ministro, ci sono anche altri scienziati, quelli che dicono che non ci sarà una seconda ondata, quelli che lavorano in silenzio, quelli che vengono derisi perché non appartengono alla linea ufficiale. allora ci dite, e lo dite agli italiani, quali sono gli scienziati i cui orientamenti mettete alla base delle vostre ragioni, oppure l'unica ragione per cui volete continuare a parlare di stato di emergenza è perché perché fa comodo a questo Governo e fa il vostro gioco che va a ricadere sulle paure degli italiani perché voi siete aggrappati alle poltrone? Siete un Governo nato nelle stanze di un palazzo, non legittimato dal voto dei cittadini, diviso su tutto, e rimanete lì soltanto grazie a questa emergenza, che tiene e funge da collante. *(Applausi)*. Voi lo sapete che le persone non si curano? Che ci sono ragazzi che hanno paura di abbracciare anche i propri nonni che non escono di casa?

È passato un mese da quando ci sono stati gli Stati generali e devo dire che, da questi, è uscito il vuoto cosmico: non c'è nulla. Non c'è un piano che dia una visione per le future generazioni; niente per i più deboli, salvo avere, forse, la proroga del divieto di licenziamento (questa, però, non è una politica per i più deboli); non ci sono politiche per le aziende: zero, assolutamente zero. Servono *leader* diversi, lungimiranti. Servono istituzioni di garanzia forti, valori e principi condivisi. Certo, il nostro bellissimo presidente del Consiglio Conte non può essere definito lungimirante, se non per il proprio tornaconto personale, non sicuramente per quello degli italiani. Così come, quando parliamo di istituzioni, il caso Palamara parla da solo. Anche qui, però, il ministro Bonafede, è ben aggrappato alla sua sedia, così come i detenuti sono tutti a casa, ben rilasciati secondo i suoi provvedimenti. Per non parlare poi della scuola, con un Ministro davvero imbarazzante che è stato commissariato da un Commissario anche lui imbarazzante, perché, comunque, è stato in ritardo su tutto.

vediamo che essi sono stati sovvertiti. Si danno priorità agli immigrati, ai *transgender* e ad altre tematiche che nulla hanno a che vedere con quei valori. Qual è l'insegnamento che date ai nostri giovani? Che cosa gli passate? Quali sono i valori e i principi della società futura? Altro che buon senso! Qui si va oltre il buon senso e il decoro! *(Applausi)*. E poi il Parlamento, che avete trasformato in un votificio.

che ci sono gli strumenti giuridici: ci sono i decreti-legge, ci sono le ordinanze contingibili e urgenti in materia di salute ed igiene. Le applichi, signor Ministro, non servono strumenti eccezionali: il nostro ordinamento ha già gli strumenti. Nella risoluzione che abbiamo presentato diamo dei suggerimenti. Vi togliamo ogni alibi nel dire che le minoranze non collaborano. Avete bocciato tutti

noi presentata vi sono dei punti chiari, così non avete l'imbarazzo di pensare a come fare le cose. Non ci sono delle limitazioni dei diritti costituzionali. Noi abbiamo a cuore la salute dei cittadini e abbiamo a cuore la loro sicurezza, senza bloccare tutta l'Italia. Per noi questo è fondamentale. signor Ministro, per non votare la nostra risoluzione e per bypassare ancora una volta il Parlamento? Potrete non rispondere oggi qui, ma lo farete di fronte agli italiani.

quindi, questo dovrebbe dirle qualcosa. Per contro, crediamo che essa corrisponda più a un desiderio del Governo prolungare di fatto uno stato di soggezione da parte di tutti i cittadini e che alla base, forse, ci sia la vostra speranza di accrescere i consensi. Le darei un consiglio, signor Ministro, anziché continuare ad incentivare l'ansia dei cittadini amplificando i pericoli (come ha fatto oggi nella sua relazione) di un'emergenza che oggi assolutamente non esiste (non lo diciamo noi, lo dicono i dati che sono noti a tutti gli italiani e che tutte le sere hanno modo di ascoltare), credo che il Governo dovrebbe assumere un atteggiamento molto più equilibrato: essere certamente capace di preservare la salute di tutti i cittadini (che sta a cuore a noi

ma quando ve ne renderete conto non vorremmo che fosse troppo tardi. Non vorremmo che questo Governo avesse lo stesso atteggiamento che ha usato nel gennaio 2020, quando tutto l'Esecutivo ha perso un mese di tempo perché voleva tranquillizzare la cittadinanza. Abbiamo visto esponenti e capi di partiti politici che venivano a Milano a fare gli aperitivi, con molti assembramenti, o sindaci di importanti città che dicevano che bisognava abbracciare i cinesi perché non c'era alcun problema. Siccome allora di tempo ne avete perso tanto, non vorremmo che adesso perdeste altro tempo non occupandovi di ciò che questa Nazione subirà a causa della pandemia - che certamente non è colpa di nessuno - da un punto di vista economico.

di controllare gli sbarchi nella nostra Nazione. *(Applausi)*. Non vi sfuggirà che i numeri sono impietosi e stanno aumentando in maniera esponenziale. Oltretutto lì non ci sono controlli lo vediamo tutti i giorni, perché sono ampiamente documentate dalla stampa tutte le fughe da questi centri di accoglienza di immigrati che dovrebbero star lì a fare la quarantena e invece vanno in giro tranquillamente, senza essere limitati in alcunché, su tutto il territorio nazionale, portando in giro il Covid-19.

per bloccare il traffico degli scafisti e l'immigrazione illegale. Non soltanto non ascolta con attenzione, Ministro, la nostra posizione è che forse è meglio non limitare le libertà individuali, ma controllare questi flussi migratori illegali che invece nessuno controlla e di cui nessuno si occupa.

con l'opposizione, una limpida dialettica tra maggioranza ed opposizione; un confronto a tutto campo, a partire dalle forze politiche presenti in Parlamento.

di Paesi e adottiamo misure che il Gruppo Italia Viva-PSI giudica proporzionate e ragionevoli, legate - come sono - al principio di temporalità. le sue motivazioni - è che nel caso della pandemia e in molti altri casi che la storia manifesta, la storia non è stata affatto - come si sostiene - *magistra vitae*, ma è stato tutto il contrario, perché soprattutto attorno a noi si sono ripetuti degli errori e delle procedure che erano decisamente note fin dall'antichità. dall'antichità. Reputiamo come fattore positivo - lo ha detto lei a conclusione della sua relazione - la concertazione fatta con il Parlamento, prevista da una norma (ma al di là della norma che la prevede), e diventata una sorta di condotta non condotta non marginale ma fissa. È una decisione convincente e vorrei che significasse - ci tornerò fra pochissimi minuti - una sorta di superamento dell'emergenza istituzionale.

Non avendo alcuna obiezione in merito, preferisco utilizzare i minuti che mi restano per cinque considerazioni. durante i mesi della pandemia abbiamo dichiarato eroi i medici e i loro assistenti per l'attività che hanno svolto. Forse ora è il caso di

Forse è venuto il momento di trattare la questione con la delicatezza e la determinazione proprie di un Paese civile, che è in grado di rileggere anche alcune regole di fronte a situazioni di crisi e di straordinaria emergenza. La seconda delle questioni: toglierei, ministro Speranza, la disposizione che ascoltiamo ormai in tutte le stazioni d'Italia, in tutti gli aeroporti d'Italia, che è sbagliata: non è distanziamento sociale, è distanziamento fisico. Utilizziamo distanziamento fisico e non sociale. In terzo luogo, aggiungo e sottolineo una parte delle considerazioni fatte da lei e poi vengo alle conclusioni; raccomando anch'io un coordinamento stretto e deciso tra le Regioni e il Governo, senza dimenticare le città. Infatti, nel corso di questi mesi le Regioni hanno lavorato costantemente col Governo, un po' meno - mi pare - i Comuni. Ma poiché le grandi città sono decisive nell'articolazione istituzionale e per le misure che si assumono, a quel tavolo deve sedere stabilmente anche l'ANCI. Infine, tre considerazioni. La prima l'ha già fatta lei e io la sottolineo con uguale forza e con maggiore determinazione: lo stato di emergenza deve essere maneggiato con cura, anzi, con moltissima cura, perché le norme eccezionali non divengano in qualche modo la norma di riferimento. Se il Governo dovesse muoversi in questo campo, perlomeno prenda in esame l'ipotesi di lavorarci con un decreto-legge, non più con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e porti le ragioni per le quali noi potremmo trovarci (uso il condizionale del verbo potere: potremmo trovarci) anche nel paradosso di avere di nuovo lo stato d'emergenza con elezioni regionali, amministrative e *referendum* convocati proprio nel corpo dell'emergenza. riguarda le scuole. Ci sono alcune misure previste nell'articolato del decreto rilancio. Il mio modello, il modello dei miei figli non è stato - forse per uno sì - il modello di Gian Burrasca, però la fisicità è parte dell'insegnamento, soprattutto nelle scuole primarie. Se non c'è fisicità la capacità e la possibilità di insegnare cadono e perdono Siccome, nonostante gli sforzi straordinari di un grande cervello (Oxford) e di una impresa piccola, ma non mediocre, italiana, romana, di Pomezia,

pare sia a un ottimo punto, ma non riusciremo ad assicurare all'Italia e agli altri Paesi la vaccinazione di massa), sapere come le scuole riapriranno diventa un fattore decisivo. Mi permetto di segnalare, in conclusione, un elemento che non è legato a un numero, anzi eviterei di citare i numeri. Io inorridisco quando sento parlare di numeri di Covid-19 in Africa; in Africa c'è un medico ogni 20.000-30.000 persone sapere quanti siano i malati o i morti di Covid-19 in Africa è assolutamente impossibile. Lo dico per sollecitare attenzione sugli sbarchi che dovessero esserci. Nella risoluzione ne facciamo riferimento: devono essere approntate misure di sicurezza e di vigilanza in quarantena che non siano gravose per le comunità.

ministri del 14 luglio è la proroga, fino al 31 luglio, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno e delle ordinanze del Ministero della salute del 30 giugno e del 9 luglio. Quindi, l'allegato contiene le nuove linee guida per le informazioni agli utenti

e ha senso prorogarle. Si tratta di ordinanze e non hanno necessità

viaggi, chiusura delle frontiere laddove necessario, *lockdown* mirati. Per tutto ciò bastano le ordinanze del Ministro della salute.

fino a dicembre, ma anche ottobre, perché si tratta, di nuovo, di un pericolo possibile e probabile, ma - appunto - di un pericolo e non di una reale emergenza. Il Ministro ha menzionato anche il vaccino, su cui vorrei soffermarmi. Avendo lavorato proprio sulla piattaforma del vaccino per più di vent'anni, voglio invitarvi

(mi permetto di parlare in questa modalità). La prima criticità è che non si sa quanto dura la risposta neutralizzante contro questo virus e, quindi, l'efficacia di un vaccino non è assicurata. Non mettiamoci in testa che torneremo alla normalità solo quando ci sarà il vaccino, perché non è detto che ci sarà un vaccino efficace e duraturo. Quanto alla seconda criticità, vedo con preoccupazione proclamare che a ottobre o in primavera avremo un vaccino. Non è così, per fare un vaccino efficace e sicuro ci vogliono almeno due o tre anni. Quindi, evitiamo deroghe alle regole normali di sperimentazione di fase 3. Dico questo anche con un invito a rispondere a un'interrogazione che ho presentato su questo argomento; sul sito del Ministero della salute si parla di terapia compassionevole per un vaccino, il che non ha senso perché un vaccino è un qualcosa che previene e che non cura. Oltre ai profili di sicurezza che la somministrazione di un vaccino può avere, in questo tipo di malattie esiste anche un altro tipo di reazione che si chiama *antibody-dependent enhancement*, che potrebbe causare maggiori pericoli a chi fa il vaccino, dando un'iperattivazione della risposta immunitaria. Dico questo per invitare a essere cauti. Io sono contentissima che dall'IRBM venga un vaccino, ma deve passare tutte le fasi di sperimentazione clinica necessarie. Occorrono due anni. A nessuno venga in mente di usarlo come terapia compassionevole, come è scritto sul sito del Ministero della salute: ciò non ha senso e ne approfitto per dirlo in questa sede. Per quanto riguarda la scuola,

insegnanti e pensare a una scuola diversa. Non voglio dire che il comitato tecnico-scientifico non sia utile - lo è - ma è poi il Parlamento che sa come deve evolvere la scuola da settembre in poi e decidere le modalità di ripresa delle attività scolastiche. Non riduciamoci a mascherine, distanziamenti e isolamenti, perché non è questa l'idea di Paese che noi, che pure abbiamo dato la fiducia a questo Governo, vogliamo sostenere. Siamo d'accordo, quindi,

emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Così è stato: limitati e predefiniti limiti

si dice che le disposizioni del decreto si applicano alla data del 15 giugno fino al 14 luglio. Si sta facendo questo fino al 31 luglio. Nessuno ha parlato di altro, nessuno ha parlato di un'emergenza ulteriore. Su questo ovviamente il Parlamento dovrà dire la sua, ma nessuno qui ha detto che stiamo andando oltre. Lo dirà il *Premier*, come lei ha detto, quando verrà in Parlamento, come noi desideriamo. Poniamo intanto l'attenzione su quello che c'è e non facciamo confusione almeno su questo, visto che i cittadini ovviamente

sappiamo che sono in corso dei monitoraggi e quindi il fatto di intervenire in emergenza per isolare questi piccoli focolai serve ovviamente ad avere dei provvedimenti adeguati.

vigilare, controllare, verificare e poi mettere in atto; dopo, sì, si potrebbe predisporre un protocollo per evitare le pandemie, ma dopo aver visto quello che è già successo. Lei, signor Ministro, ha dato comunque anche ulteriori indicazioni, che ha citato (vaccino;

con la dialettica che ci dev'essere fra Governo e Parlamento, dobbiamo andare avanti su questa strada, senza abbassare la guardia, perché - come abbiamo già visto - il virus non è scomparso. Dobbiamo stare attenti

di scienza conosco meno di quanto sarebbe necessario. Anche per questo, ma non solo, non entro nella disputa tra rigoristi e negazionisti che sta attraversando il nostro mondo scientifico. So qualcosa però di metodologia delle scienze sociali e allora, signor Ministro, mi permetta di correggerla su questo: il rischio zero non esiste.

che abbiamo vissuto un'esperienza e che oggi non ci troviamo più in quella situazione. Signor Ministro, l'Italia vive nel mondo in cui vivono anche gli altri Paesi occidentali: il Belgio ha fatto cessare l'emergenza il 30 giugno; Cipro il 17 maggio; la Repubblica Ceca il 14 maggio; l'Estonia il 17 maggio; la Finlandia il 15 giugno; l'Ungheria il 16 giugno; la Lettonia il 9 giugno; il Lussemburgo il 24 giugno; la Romania il 15 maggio; la Slovacchia il 12 giugno; la Spagna il 21 giugno; la Lituania il 10 giugno; Malta il 16 giugno; la Polonia il 2 giugno; la Francia ha fissato il più incosciente di noi; probabilmente c'è un idea dell' emergenza che è più simile a quella che io ho identificato, piuttosto che a quella che ho colto dalle sue parole. Che cosa è legato a un'eventuale proroga dello stato di emergenza? Signor Ministro, io colgo due conseguenze ed entrambe - devo dire la verità - mi fanno un po' paura. Una dal punto di vista istituzionale:

ministri abbiamo in alcuni casi inciso anche su libertà costituzionali. Perfino le FAQ pubblicate sul sito di un Ministero hanno avuto forza legislativa in un momento di emergenza. Signor Ministro, le ripeto: i suoi studi sono abbastanza approfonditi e lei sa che nel nostro ordinamento ci sono i decreti-legge che sono provvedimenti di necessità e di urgenza. Essi sono stati e vengono ancora usati in maniera impropria da tutti i Governi, di destra, di sinistra, di centro, per cercare di andare avanti. E invece una volta che la necessità e l'urgenza ci sono veramente, questo strumento lo prendiamo e lo mettiamo da parte. Lei ha fatto una forte perorazione a favore del Parlamento; l'unico modo di tradurla in fatti è ripristinare la gerarchia delle fonti e restituire al Parlamento quanto meno un ruolo di controllo.

«Spillover» di Quammen e sono arrivato alla conclusione che noi abbiamo sottovalutato per molti anni le pandemie, indipendentemente dal coronavirus. E se dobbiamo imparare qualcosa da ciò che abbiamo vissuto è che la vera emergenza è quella di cambiare la nostra normalità e in qualche modo di governare quello che è accaduto in questi mesi, anche se, secondo la sua concezione, arrivassimo al rischio zero. Noi non possiamo più stare in Parlamento nello stesso modo; non possiamo più andare a lavorare nello stesso modo; non potremo più stare a scuola nello stesso modo; non potremo andare in uno stadio di calcio allo stesso modo. Ciò che dunque dobbiamo fare è governare il cambiamento, rendendolo compatibile con la sostenibilità economica. Questa è la vera sfida emergenziale che abbiamo davanti. Però, per fare questo, è necessaria una visione. Io spero che il Governo ce la comunichi e che non ci dica, nei fatti, che la sua unica visione è l'emergenza. *(Applausi).*

Signor Presidente, ci pare che il Governo abbia finalità diverse da quelle dichiarate. Si vuol far passare per comunicazioni su misure di contenimento del dei ministri che è l'anticamera per giustificare il preannunciato prolungamento delle misure estreme di emergenza nazionale. Ora, è di tutta evidenza che il virus oggi viene approcciato in modo assolutamente diverso, soprattutto per tempestività di tracciamento e di diagnosi precoce, che non erano assolutamente standardizzati all'inizio dell'epidemia. Quindi fortunatamente, non sarà replicabile lo *stress test* a cui è stato sottoposto il nostro sistema sanitario in marzo-aprile. Quello che invece manca è un vero sistema di prevenzione pandemica nazionale, sorveglianza, controllo e profilassi internazionale a cui il Governo ha fatto orecchie da mercante, trasferendo la catena delle responsabilità a livello territoriale,

un piano antipandemia, che quantomeno oggi dovrebbe arricchirsi delle recentissime esperienze e delle crescenti conoscenze cliniche, farmacologiche organizzative, ma, in quanto proveniente da un'opposizione sgradita, non viene nemmeno preso in considerazione; mentre invece, con la sua pronta adozione, si andrebbero a risolvere gli innumerevoli *vulnus* strutturali che hanno contribuito all'acuirsi della crisi economica. Sarebbe sufficiente, per quanto riguarda il versante sanitario, la realizzazione di una centrale nazionale delle emergenze (sul modello CDC), delegando a competenze e conoscenze già presenti presso il Ministero della salute, come il Centro controllo malattie, con una cabina di regia al vertice integrata dall'Istituto superiore di sanità e da una rappresentanza qualificata Stato-Regioni. Qualora si dovesse ripresentare una recrudescenza epidemica (ipotesi tutt'altro che remota), potrà dare indicazioni tempestive e prescrittive alla Protezione civile sulle azioni da intraprendere e sugli strumenti da utilizzare. Tutto questo sulla base di un aggiornato piano pandemico di prevenzione e controllo pandemico, che di fatto è una lacuna che avrebbe potuto essere già colmata in sede di conversione del decreto-legge n. atto ad escludere qualsivoglia necessità di ricorrere per la stessa fattispecie allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, che non dovrebbe attenere alle emergenze sanitarie, soprattutto e ancor di più in questo caso, posto che si tratterebbe di un su qualcosa di inedito e di storicamente unico è giustificabile che eccezionalmente decida il Governo, di una fattispecie non solo già nota, ma oggi qualificabile a bassa criticità, è più che sufficiente che se ne occupi un organismo tecnico e che le prerogative fondamentali sulle libertà costituzionali siano oggetto di attenta salvaguardia, vengano in sostanza salvaguardate dal rischio di possibili arbitrarie distorsioni. si continua a disattendere una *governance* nazionale di controllo e prevenzione pandemica, alla base di qualsiasi programma di rinnovo e di adeguamento del sistema sanitario in chiave anti e post-Covid, per un corretto bilanciamento in prevenzione, in medicina territoriale ed ospedaliera, mediante correzioni sulle regole generali di ingaggio e attualizzazione della rete,

di informazione, educazione, prevenzione, assistenza e cura delle malattie infettive e per l'adoperarsi di quanto è necessario affinché l'eventualità di una nuova ondata pandemica non abbia ulteriori effetti avversi. Emergenze come quella del Covid hanno fatto male, e se non si pone rimedio ne faranno sempre di più, a chi è più fragile, non solo sotto il profilo sanitario e socio-sanitario, ma economico e sociale. Invece che misure assistenzialistiche destinate a esaurirsi improduttivamente, occorre agire da subito in prevenzione pandemica, quale leva fondamentale per il contrasto delle vulnerabilità sociali ed economiche, precondizione del benessere individuale e collettivo e presupposto ineludibile per il superamento dell'emergenza economica che stiamo vivendo

Signor Presidente, colleghe e colleghi, gentile Ministro, la ringrazio per la sua così esaustiva relazione che ha illustrato chiaramente perché la proroga delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno sia un atto doveroso. Ho l'impressione che nel Paese si stia diffondendo l'errata opinione che l'emergenza sia finita e ci si stia dimenticando di quello che è stato. stato. Permettetemi quindi di ricordare in quest'Aula alcuni dati estrapolati dal rapporto dell'Istat denominato «Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel primo trimestre 2020». Considerando il solo mese di marzo, a livello medio nazionale si osserva una crescita del 49,4 per cento dei decessi per il complesso delle cause; se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid (il 20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi passano da 65.592, che è la media del periodo 2015-2019, a 90.946 nel 2020. L'eccesso dei decessi a livello nazionale è di 25.354 unità. A causa della forte concentrazione del fenomeno in alcune aree del Paese, i dati riferiti al livello medio nazionale appiattiscono la dimensione dell'impatto dell'epidemia di Covid sulla mortalità totale. Il 91 per cento dell'eccesso di mortalità riscontrata a livello medio nazionale nel mese di marzo 2020 si concentra nelle aree ad alta diffusione dell'epidemia, circa 3.000 Comuni in 37 Province del Nord più Pesaro e Urbino. Nell'insieme di queste Provincie i decessi per il complesso delle cause sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015/2019 del mese di marzo. Se si considera il periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, i decessi sono passati da 26.218 a 49.351, oltre 23.000 in più. All'interno di questo raggruppamento, le Province più colpite dall'epidemia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane, con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al periodo precedente, a tre cifre.

Nelle aree di media o bassa diffusione gli incrementi sono stati decisamente inferiori. Tra questi ce ne sono alcuni per i quali non è accertata la mortalità per Covid ma è altamente possibile che vi sia un collegamento indiretto con il Covid o, infine, che una quota di mortalità indiretta non sia correlata direttamente al virus ma sia stata causata dalla crisi del sistema ospedaliero e dal timore di recarsi in ospedale nelle aree maggiormente affette dal virus. Mi auguro che questi numeri servano a dissipare definitivamente i dubbi che ogni tanto qualche sedicente medico accampa su Internet rispetto alla pericolosità del Covid e all'effettiva mortalità. È stata veramente una tragedia di proporzioni mai viste in Italia, non dobbiamo dimenticarlo e non dobbiamo abbassare la guardia. Ad oggi, in Italia si contano 243.344 casi e 34.948 morti. Nel mondo sono oltre 13 milioni i casi confermati e quasi 600.000 i morti. I casi, in questi ultimi giorni, stanno salendo al ritmo di oltre 200.000 al giorno. Anche in Italia abbiamo nuovi focolai laddove calano le misure di sicurezza: nelle nostre imprese, tra i nostri lavoratori, in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna tra persone prevalentemente provenienti in maniera regolare da Paesi esteri. Questo dovrebbe farci capire chiaramente che il virus non ha perso forza, non è meno aggressivo. È stato il nostro Governo a mettere in atto le misure giuste per fronteggiare l'emergenza, come ha ribadito anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. A marzo Italia e Spagna erano l'epicentro della pandemia di Covid. Al culmine dell'epidemia, l'Italia contava più di 6.500 nuovi casi al giorno. Il Paese ha riportato la situazione sotto controllo con una combinazione di *leadership*, umiltà, partecipazione attiva di ogni membro della società e un approccio globale. È stata affrontata una situazione spaventosa ma è stata ribaltata. Insomma, è sotto gli occhi di tutti che l'emergenza dal punto di vista sanitario a livello globale non è finita, come ha detto anche lei, signor Ministro. In Italia siamo in una fase di convivenza con il virus ma sono certa che sapremo tutti insieme scegliere le misure adatte a fronteggiarlo in maniera adeguata nei prossimi mesi. Le conoscenze sulla patologia sono aumentate e abbiamo messo in atto tutte le misure per fronteggiare un'eventuale recrudescenza dell'epidemia. Abbiamo potenziato il nostro Servizio sanitario nazionale, aumentato stabilmente il personale sanitario, quel personale a cui deve andare e a cui va tutta la nostra gratitudine per quanto fatto fino ad ora. Possiamo e dobbiamo potenziare la diagnosi precoce, soprattutto per coloro che arrivano dall'estero, attraverso una maggiore diffusione di test sierologici e molecolari, si spera i più rapidi possibile. Dobbiamo tenere il passo con l'innovazione scientifica e tecnologica, mai come in questo momento. Solo in questo modo potremo pensare, nell'immediato futuro, di poter porre termine alle poche limitazioni che ancora ci sono ma che sono indispensabili per tutelare tutti noi e contenere il più possibile il rischio

per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Schede bianche | 10 | | Schede nulle | 13 | Proclamo eletti Agostino Ghiglia, con 123 voti, e Pasquale Stanzione, con 121 voti.

il Ministro della salute, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Signor Presidente, replicherò in pochissimi minuti. Intanto, desidero esprimere gratitudine a tutte le senatrici e i senatori che hanno voluto intervenire e portare il loro contributo a questa utile discussione. Mi pare evidente che ci sia una condivisione di fondo su un punto: è evidente che il Paese è in una fase nuova ed in una fase diversa. Io ho provato a usare queste parole: siamo fuori dalla tempesta, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Questo significa che i sacrifici enormi svolti dai nostri cittadini, le misure rigorose che il Governo nazionale e le Regioni hanno assunto ci hanno consentito di superare la fase più difficile, ma è evidente che ancora non siamo in sicurezza e che abbiamo bisogno del massimo livello di cautela possibile. L'argomento, la questione, che più in questa fase ci preoccupa, evidentemente, è il quadro mondiale. infatti, questa analisi è giusta e corretta per l'Italia, se questa analisi è giusta e corretta per l'Europa, non lo è sicuramente sul piano mondiale, dove le cose peggiorano settimana dopo settimana e siamo sostanzialmente nel momento di massima impennata di questa curva.

questa battaglia chiusa e che dovremo continuare ad avere un livello molto alto di attenzione. Le misure che restano attive sono alcune delle misure essenziali, oltre a quelle che riguardano chiaramente il controllo e le questioni di monitoraggio per gli arrivi e gli accessi dei Paesi stranieri e io farò tutto il possibile perché questo avvenga nel massimo rigore. Ad oggi c'è una lista di divieti di ingresso e di transito, addirittura, per 13 Paesi e c'è la quarantena per tutti gli arrivi dai Paesi extra-Schengen ed extra-UE, ma è del tutto evidente che ci sono tre regole fondamentali che dobbiamo assolutamente chiedere ai nostri cittadini di mantenere ancora. Sono tre regole che restano i principi cardine essenziali. l'utilizzo delle mascherine e dei dispositivi di protezione e il distanziamento di almeno un metro. A tale riguardo, condivido l'indicazione che arrivava di non la dizione «distanziamento sociale»: si tratta di un distanziamento fisico di almeno un metro, che però è veramente importante. La terza regola è l'utilizzo delle misure igieniche fondamentali, a partire dal lavaggio delle mani. Questi tre restano essenziali, sono le tre armi decisive per provare ad affrontare la fase della convivenza. Anche qui - lo ripeto solo per un istante - credo che non dobbiamo commettere l'errore l'errore di porre in contraddizione la questione sanitaria con la questione economica e sociale. La penso esattamente all'opposto: ritengo che la vittoria sanitaria sia la premessa fondamentale per la ripartenza economica e sociale. Non basteranno provvedimenti o interventi di natura nazionale, internazionale, regionale, gli sforzi che pure si stanno facendo, se non avremo la capacità di tenere sotto controllo il virus. Non mettiamole in contraddizione l'una con l'altra, quindi: sono due pezzi di una strategia che dobbiamo assolutamente provare a tenere insieme. Sulla vicenda dello stato di emergenza credo di aver usato parole di grande chiarezza: nessuna decisione è stata assunta. ritengo indispensabile il confronto con il Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri sarà qui entro la scadenza dello stato di emergenza, prevista per la fine di questo mese, e avrà modo chiaramente di esplicitare un confronto vero, serrato.

di rispettare l'articolo 32 della Costituzione, quindi di difendere la tutela della salute, e al tempo stesso il bisogno di rispettare fino in fondo le prerogative del Parlamento, le fonti primarie e il nostro impianto democratico. fatemi ripetere solo per un istante un concetto che ho toccato velocemente nella mia introduzione, ma che mi sembra particolarmente significativo: all'inizio di questa epidemia, quando vedevamo le immagini della Cina e le misure incredibili che in quel Paese venivano assunte, tanti commentatori hanno segnalato come sarebbe stato impossibile, in un Paese delle libertà, in un Paese della democrazia e della tutela dei diritti individuali portata giustamente all'ennesima potenza, gestire l'emergenza. penso che la storia abbia dimostrato esattamente l'opposto. La mia opinione è che la democrazia è stata un punto di forza. Non abbiamo piegato quella curva di misure di natura securitaria che abbiamo imposto al Paese; abbiamo piegato quella curva perché siamo riusciti a costruire una sintonia profonda con i cittadini di questo Paese, che a un certo punto hanno colto fino in fondo il rischio che si correva e si sono sostanzialmente messi in uno spirito assolutamente responsabile di collaborazione rispetto alle misure che a livello nazionale come a livello regionale venivano messe in campo. quindi che dobbiamo lavorare per costruire questo equilibrio; la mia opinione è che le condizioni ci siano tutte. Come ho detto, continueremo a lavorare su alcuni punti essenziali. Ho parlato dei vaccini: è evidente che il vaccino per noi è un orizzonte da coltivare con grandissima convinzione, e vedere che l'Italia è a testa alta dentro questa partita, anche con competenze e conoscenze, con attività industriali di primissimo piano che vengono riconosciute dai nostri interlocutori internazionali, va sicuramente nella direzione giusta. Compito delle istituzioni sarà evidentemente verificare la sicurezza e fare tutto quello che è necessario perché il vaccino arrivi certamente nel più breve tempo possibile, ma nell'assoluta sicurezza. sicurezza. Da ultimo, mi sia consentito un messaggio legato più in generale al nostro Servizio sanitario nazionale. Vorrei che il Parlamento su questo fosse unito, e mi sembra che gli interventi di oggi segnalino una necessità univoca di ricominciare ad investire, di chiudere la stagione dei tagli che ci siamo portati per troppo tempo negli ultimi anni e di riconoscere nel Servizio sanitario nazionale un bene collettivo del nostro Paese, un *asset* strategico fondamentale su cui fare il miglior investimento possibile. Sono orgoglioso del nostro Servizio sanitario nazionale e sono orgoglioso in modo particolare dell'impianto e del principio universalista che lo ha ispirato e che ha messo in campo: l'idea che di fronte a un essere umano malato non deve contare nulla se non la necessità assoluta di rispondere a quel bisogno e a quelle esigenze.

parere favorevole sulla risoluzione di maggioranza e non posso esprimere parere favorevole sulle risoluzioni presentate dai senatori di minoranza, anche perché vanno molto oltre quello che è l'ambito della nostra discussione, cioè quanto indicato dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Tuttavia, voglio utilizzare questi ultimi secondi della mia replica in Senato per dire che ho letto con attenzione l'interrogazione che il senatore Romeo ha voluto rivolgermi e di cui sono soltanto ora venuto a conoscenza: mi sembra che ponga un tema di assoluto buonsenso su cui sin da subito mi impegno ad interloquire. Ritengo che il Parlamento sul tema del piano pandemico debba necessariamente essere coinvolto e che si possa costruire

perché la chiusura della stagione dei tagli - come lei l'ha definita - non è stata oggetto di una decisione politica, di una maggioranza che ha deciso di tornare ad investire nel Servizio sanitario nazionale è stata semplicemente il frutto di quello che è accaduto, cioè una delle più grandi emergenze della storia repubblicana, e necessitata evidentemente dai gravi ritardi manifestati dal nostro Servizio sanitario nazionale.

una linea di non ritorno: qualcosa che ci induce a non ripetere tutto ciò che è accaduto. Questo non lo diciamo perché vogliamo anticipare quelli che saranno i giudizi sull'attività di Governo nell'affrontare l'emergenza pandemica, ma perché è del tutto evidente che di fronte ad alcune cose magari ben fatte, molte ascrivibili agli operatori e ai volontari del nostro Servizio sanitario nazionale, sono stati compiuti leggerezze, ritardi e omissioni che evidentemente non sono auspicabili per i prossimi mesi. Soprattutto non sono ripetibili le semplificazioni, le scorciatoie, le conferenze stampa reiterate, le *fake news* diramate a reti unificate e le normative secondarie assurte a norma primaria per limitare i diritti costituzionalmente garantiti. della forma (ma vorrei dire banalmente che nelle istituzioni la forma notoriamente è sostanza, Ministro), non deve più ripetersi. Rispetto a questa vicenda io sono

una legge, che stabilisce cosa accade nel nostro ordinamento. Lettera 150 - che lei, Ministro, evidentemente conosce: sono 150 costituzionalisti che si sono impegnati nelle vicende di questa emergenza e del *lockdown* - ha espressamente confermato che sono necessari interventi, anche urgenti, magari anche attraverso decreti-legge, ma riconducibili alla ordinaria gestione legislativa parlamentare. In altri termini, in questo momento «è venuta meno (...) quella condizione che ha permesso, sino ad oggi, la sospensione di diritti costituzionali fondamentali. Lo stato di emergenza, infatti, è una grave circostanza imprevista che richiede misure immediate di intervento, non compatibili con i normali tempi di elaborazione e proclamazione di leggi e provvedimenti amministrativi ordinari». «La sola idea che una proroga dello stato di emergenza possa non essere deliberata dal Parlamento, e anzi gli possa essere sottoposta solo per un "passaggio" dal contenuto e dalle finalità incomprensibili, è inconciliabile con il nostro ordinamento costituzionale». Segue una serie di altre considerazioni. Questo è il senso del ragionamento sul quale noi oggi ci dobbiamo soffermare ed esprimere, Ministro: o e allora si aprono scenari di un certo tipo, oppure questo virus, come dicono purtroppo in tanti, non c'è o perlomeno non c'è più come era o perlomeno non è più così letale come era all'inizio,

invece essere prodotti provvedimenti mirati, sì, ma attraverso gli strumenti previsti dal nostro ordinamento, della nostra gerarchia di fonti e i provvedimenti, evidentemente, devono essere mirati alla bisogna e quindi anche territorialmente, oltre che temporalmente, circoscritti. Dopo di che, vanno anche protette le frontiere, Ministro. Lei ha giustamente detto che proteggeremo le frontiere non io le suggerisco, Ministro, di dare un'occhiata anche alle frontiere europee, perché, nella mia Umbria, gli ultimi cinque contagiati sono, casualmente, cinque badanti, che stavano dentro un pulmino che veniva dal Nord Europa: sono state tutte asintomatiche,

da quei Paesi. Oppure c'è l'altra ipotesi che io considero, Ministro, e che condivido: il virus c'è; forse è cambiato, forse è intervenuto il caldo, forse semplicemente abbiamo cambiato i protocolli di cura - finalmente, aggiungo - e quindi è meno aggressivo, meno virulento,

udite bene: un ordine del giorno unitario, che meriterebbe una sorta di monumento fuori dall'Aula del Senato - contenente sette impegni. lei era presente in Aula. Questi sette impegni, che non leggo perché non ho tempo, sono tutti importanti se il virus c'è: ripeto, sono assolutamente importanti perché attengono alla capacità di trovarlo, scovarlo, curarlo, isolarlo e risolverlo.

l'indagine di sieroprevalenza è fallita e se ne sono perse le tracce, anzi, i test sierologici sono scaduti

Come ho detto, l'indagine di sieroprevalenza ha prodotto risultati modesti, anzi impercettibili. In ogni caso, Ministro, dobbiamo agire con una chiarezza di intenti. Nelle due strade - o l'una, o l'altra - prendetevi la responsabilità di dirci che cosa accadrà. E non potete farlo con la proroga dello stato di emergenza (cioè, in poche parole, per chi sa giocare a tressette, come: passa). Non è così che si governa. C'è bisogno di una visione, di una previsione e di una strada tracciata. Mi rendo conto che questo è un Governo che fatica a trovare l'alchimia della

strumenti messi a disposizione dei legislatori - cioè l'uso del decreto-legge o della fiducia

parlamentare. Signor Ministro, lei oggi ha detto una cosa che condivido appieno, cioè che non basta una comunicazione, seppur fatta autorevolmente dal Presidente del Consiglio, di proroga dell'emergenza al 31 dicembre

Credo che abbiamo bisogno della garanzia da parte sua e da parte del Governo che qualunque tipo di provvedimento sul tema dell'emergenza dell'emergenza abbia un passaggio parlamentare vero e soprattutto dobbiamo riuscire a garantire percorsi che facciano sì che trasmettiamo messaggi diversi al Paese rispetto a quelli che abbiamo trasmesso finora, signor Ministro, la fase è cambiata, è mutata profondamente rispetto a prima. Sono convinto che sia corretto che il Ministro della salute intervenga qui in Parlamento per dire che dobbiamo tenere alta la guardia;

commetteremmo un errore se pensassimo che soltanto di questo oggi dobbiamo occuparci. Ricordo, ad esempio, che lei qui oggi è presente come delegato del Presidente del Consiglio rispetto alle comunicazioni che si fanno in Parlamento,

però che oggi sarebbe stato un segnale interessante, proprio per dare il senso del cambio di marcia rispetto a quello che abbiamo gestito fino ad ora, che insieme a lei o addirittura al posto suo, delegato per il Presidente il Consiglio potesse essere il ministro Patuanelli o il ministro Gualtieri, proprio perché oggi, seppur con l'atteggiamento di chi deve tenere alta la guardia, dobbiamo capire quali provvedimenti mettere in campo, prendendo atto che la fase è mutata e quindi dobbiamo comprendere come non sosteniamo più soltanto con misure assistenziali l'economia di questo Paese, non ci preoccupiamo più soltanto dell'emergenza sanitaria, che per fortuna attualmente è superata. Diciamolo, Ministro: in questo momento l'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato qualche settimana fa, per fortuna, nel nostro Paese è superata. Non bisogna ricascarci, bisogna essere pronti ad arginare eventuali altri focolai, ma è superata e se continuiamo a giocare la stessa partita che giocavamo quando eravamo in piena emergenza, commettiamo un errore. Per questo è sbagliato, anche soltanto in una conferenza stampa, anticipare una proroga al 31 dicembre delle procedure di emergenza e di gestione dell'emergenza sanitaria di questo Paese. Dobbiamo, semmai, dare un segnale diverso al Paese. Se la classe politica, le istituzioni e il Governo continuano a dare segnali difensivi, cosa devono pensare i cittadini? Come devono comportarsi? Credo che da questo punto di vista ancora non abbiamo marcatamente segnato la differenza tra una fase e l'altra e credo che il Governo abbia delle responsabilità precise nel manifestare questo cambio di guardia, di atteggiamento. Lo dico perché abbiamo misure eccezionali, in materia economica, da mettere in campo e dobbiamo anche evitare di essere contraddittori in materia sanitaria, Ministro. Non possiamo dire che c'è l'emergenza, fare l'elenco delle cose che lei ha detto e che io condivido e dopodiché, ad esempio, non prendere in emergenza le risorse del MES, perché o l'emergenza sanitaria c'è e quindi abbiamo bisogno di risorse straordinarie rispetto alla gestione del nostro sistema sanitario, oppure possiamo farne a meno perché il nostro sistema sanitario regge e non c'è bisogno di risorse che ci vengono messe a disposizione dall'Europa per fare assunzioni tra i medici e tra gli infermieri, per migliorare la medicina territoriale, per migliorare le nostre strutture sanitarie, per migliorare tutto ciò che riguarda le terapie intensive. Delle due l'una, ma le due azioni insieme, una contraddittoria rispetto all'altra, non vanno. Credo quindi che da un lato dobbiamo cambiare totalmente e radicalmente verso rispetto alle misure che dobbiamo prendere in materia economica, sfruttando appieno le risorse che speriamo presto ci metterà a disposizione l'Europa. Ricordo che in grossissima parte abbiamo speso gli 80 miliardi

che ci separano dalle prossime comunicazioni del Presidente del Consiglio, anche con i Ministri economici, perché il primo cambiamento che dobbiamo manifestare nei confronti degli italiani è che ci stiamo preoccupando della vera emergenza attuale, che è quella economica. Sono convinto, come dice lei, che le due questioni non vadano in contraddizione, però in questo momento cambiano le priorità: sia alta la guardia - ho sentito il senatore Romeo proporre un elenco di

e personaggio da citare rispetto a chi sostiene che Conte sta prendendo i pieni poteri; mi sembra veramente incredibile che chi ha aspirato ai nuovi poteri possa oggi dire che Cassese è diventato il suo punto di riferimento.

cambiare verso, dando un ruolo maggiore al Parlamento e alle istituzioni democratiche. Noi non staremo lì, signor Ministro, ad ascoltare silenti eventuali provvedimenti di chiusura del Paese, con proroga delle condizioni di emergenza al 31 dicembre, senza che vi sia stato un coinvolgimento della maggioranza, dell'opposizione e del Parlamento. Credo che su queste misure ci sia bisogno di un coinvolgimento di tutti, che sia possibile mettere in campo azioni che risollevino finalmente il Paese con misure economiche straordinarie e che, al tempo stesso, si possano garantire sicurezza sanitaria, distanziamenti e tutto quello che ha citato, senza però continuare a mettere questa come azione prioritaria, mentre il Paese chiede aiuto rispetto alle misure economiche. Altrimenti, signor Ministro, quando scadrà

essere inondati da licenziamenti. Per me la proprietà oggi è quella e vorrei che il Governo se ne occupasse, pronto ad arginare qualunque emergenza sanitaria, ma prontissimo a rimuovere tutti gli ostacoli che ci separano da un rilancio economico complessivo.

con onestà intellettuale, possiamo riconoscere un primo punto su cui ritrovarci: ciò ciò che è accaduto nei mesi che ci stanno alle spalle era inedito, nessuno era «imparato», e non c'è dubbio che le azioni messe in atto dal Governo e dalle Regioni abbiano dimostrato un'efficacia, almeno per limitare, governare e convivere, come abbiamo avuto modo di dire tante volte in quest'Aula, con

non perché dobbiamo sottovalutare i limiti e i problemi veri che abbiamo incontrato in questi mesi, ma perché, se guardiamo al panorama mondiale, è evidente che l'Italia, primo Paese in Occidente ad aver dovuto fare i conti con il coronavirus, abbia retto in modo diverso e sostanzialmente migliore rispetto ad altri Paesi, e non solo a Paesi arretrati ma anche avanzati (penso ad esempio agli Stati Uniti). La cosa ci dovrebbe consentire - non è adesso il momento - di fare una riflessione più complessiva sui modelli sanitari

non continuiamo nella retorica, per me abbastanza stucchevole, degli eroi e magari pensiamo strategicamente a riconoscere loro, contrattualmente, ciò che è giusto riconoscere. È merito delle istituzioni locali ed è merito degli italiani. Noi qui - dico «noi» perché non voglio fare assolutamente polemiche - abbiamo ascoltato a più riprese andamenti molto ondivaghi rispetto al tema del coronavirus. Gli italiani

Ora, colleghi, dire questo, che mi sembra un ragionamento di onestà intellettuale, significa sottovalutare i problemi i drammi che dal punto di vista economico e sociale stiamo vivendo e vivremo nei prossimi mesi? Assolutamente no. Assolutamente no. Non credo che qui abbiamo bisogno di fare la gara tra chi è più preoccupato della situazione economica e sociale; ne siamo tutti convinti e stiamo e dobbiamo cercare di fare di più e meglio. L'unica cosa che non possiamo fare è contrapporre questo ragionamento al tema della

Dunque, noi oggi ci esprimiamo su una proposta che ci avanza il Governo e cioè un aggiornamento del decreto del Dobbiamo confermare il distanziamento. Io sono d'accordissimo e l'ho proposto anche in un precedente dibattito: non il distanziamento sociale, ma il distanziamento fisico.

Condivido - e lo dico senza incertezze, anche ai colleghi dell'opposizione - che bisogna fare la massima attenzione e avere la massima garanzia,

per i Paesi extra-Schengen e, tanto più, per le situazioni di emergenza come quella appunto degli sbarchi. Non c'è ragione, da questo punto di vista, di dividerci tra noi, perché questa è la scelta giusta che dobbiamo fare. Oggi poi si è aperta un'altra discussione, che non è oggetto di questo dibattito e che attiene al tema

Non mi capita spesso di essere d'accordo e di citare il senatore Faraone, tuttavia un po' meno comunicazione su questo punto, prima di aver deciso, preso un orientamento e coinvolto il Parlamento, sarebbe ed è una cosa utile. Infatti di "annuncite" dobbiamo riuscire a fare a meno in questo Paese. Secondo me questo è molto importante. Però, colleghi, la risposta che ha dato il Ministro è una risposta seria: verrà il Presidente del Consiglio e discuteremo nel merito, anche del tipo di provvedimento. Io dico che ci sono le condizioni per ragionare sul tipo di provvedimento. Ma l'idea

sarebbe legata a un tema di tutela del Governo francamente è un'ipotesi che non fa onore all'intelligenza di chi propone questo ragionamento. ragionamento. In verità noi dobbiamo avere un attenzione perfino culturale. Il Paese ha reagito bene e dobbiamo evitare che passi l'idea il problema è risolto; dobbiamo invece trovare quelle articolazioni e quegli equilibri per evitare che il Paese "pendolarmente" discuta di chiusure e di *lockdown* totale o di liberi Ci sono altre strade normative e perfino altri percorsi parlamentari, magari sulla base di un impegno sui tempi da parte di tutte le forze politiche che stanno in Parlamento (Camera e Senato), per vedere per vedere se si riesce a trovare l'equilibrio giusto a garanzia delle due necessità che abbiamo di fronte. Ho finito il tempo, per cui

Ma riorganizzazione, ridefinizione e rivalutazione anche del modo in cui possiamo gestire, da qui a dieci anni, l'evoluzione tecnologica e scientifica che attraversa la sanità. Voglio solo ancora una volta sottolineare un punto: la scuola. Signor Ministro, lei lo ha posto giustamente come un punto centrale lo voglio dire in termini molto chiari: dobbiamo riaprire le scuole in sicurezza e non pensare a scorciatoie che non possono reggere. Scuole in presenza. Il Governo deve mettere a disposizione ulteriori provvedimenti straordinari per l'assunzione di insegnanti e per strutture e aule dove sia possibile fare formazione scolastica in presenza; tutto il resto è solo confusione e, come ho già avuto modo di dire, gli italiani su questo punto non ci perdonerebbero.

a seguire l'evoluzione della pandemia nel nostro Paese e anche a ripetere parole che sono la dimostrazione del fatto che non siamo usciti da questa situazione, non siamo usciti dalla pandemia, siamo ancora in una condizione che ci obbliga a tenere alta l'attenzione nei confronti del virus.

rappresentino una risposta che ha ancora un senso, un significato, un'importanza, ma che non rappresenta più il tutto

prepariamoci a fare in modo che una seconda ondata non ci colga impreparati, ma ci dia la possibilità di dare una risposta significativa, tempestiva, positiva. ci sono le risorse per intervenire sul nostro sistema sanitario e dare una risposta incisiva ad un ritorno del virus che fosse che fosse significativo, imprevedibile. Ci auguriamo ancora che non ci sia questo ritorno del virus, però lì abbiamo messo le risorse, abbiamo costruito le azioni per non essere impreparati.

avviso alcuni aspetti che oggi venivano anche ricordati in altri interventi debbono avere e trovare delle risposte e delle riflessioni più approfondite. conto, infatti, è mettere in campo le risorse per affrontare l'emergenza, un conto è dare progettualità per uno sviluppo, per una dinamica di modificazione del sistema sanitario nel nostro Paese.

se a livello di emergenza sanitaria e di misure di emergenza possiamo scegliere di investire sul territorio con le unità speciali di continuità assistenziale a livello di azioni di emergenza possiamo investire assumendo nuovi medici, infermieri e OSS, costruendo presidi anche attraverso l'istituzione dell'infermiere di comunità, se, nel momento in cui dobbiamo affrontare l'emergenza, le azioni sono concentrate sugli investimenti, sui Covid hospital - anche queste sono misure specifiche quali le Regioni hanno fatto le loro valutazioni e, come ci ha detto il Ministro, si è arrivati ormai in fondo alla valutazione di tutti gli investimenti che devono essere fatti - dopo sarà il problema dell'omogeneità del Servizio sanitario sul territorio nazionale che, essendo composto da sanità regionali, non ha oggi regionali, non ha oggi la prospettiva di un percorso di convergenza. La progettualità deve andare in questa direzione.

tra i vari livelli istituzionali, ma è quello che dobbiamo fare se veramente vogliamo traghettare la sanità, in termini di investimenti e di nuovi livelli di servizio omogenei a livello nazionale e quindi sui vari territori, per uscire

recepito dalle varie Regioni. Le Regioni lo hanno recepito secondo i modelli sanitari che stanno applicando, quindi in modo assolutamente differente. Rispetto a questo, il tema delle cronicità, che purtroppo abbiamo incontrato nel corso della pandemia, è un piccolo esempio significativo di come dobbiamo andare verso una convergenza dei sistemi sanitari regionali.

qualcosa di conosciuto, una prospettiva che ci si senta in grado di affrontare, un pezzo di futuro che riguarda la propria vita che le condizioni e il contesto consentano di affrontare con fiducia.

soprattutto economica e sociale, sono nel *green new deal* e in alcune parole d'ordine che devono rappresentare obiettivi ma anche strade concrete per le nostre imprese, per le nostre famiglie, per i nostri cittadini, per i nostri lavoratori. Questo dobbiamo costruire. Perché, se è vero che siamo di fronte a un terzo dopoguerra, questa volta non ci sono da ricostruire delle strade e dei palazzi, ma c'è da ricostruire la comunità. E la comunità si costruisce dando fiducia e costruendo solidarietà. Io ritengo che questo sia il nostro obiettivo e questo ritengo sia l'elemento che dobbiamo costruire attraverso le azioni che verranno. Azioni che, a mio parere, dovremo valutare, insieme con il Presidente del Consiglio, insieme con il Governo, in quale modo e attraverso quali strumenti sarà più opportuno attuare. Secondo me, vi sono delle azioni di tipo economico che abbiamo potuto mettere in campo perché c'era lo stato di emergenza. In una condizione normale, non credo si possano obbligare le aziende a non licenziare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, nei giorni scorsi il Presidente del Senato ha dovuto lanciare un grido d'allarme, parlando di un Parlamento, di un Senato, diventato una sorta di luogo degli invisibili; un grido d'allarme che, francamente, condivido, perché in molte occasioni il Parlamento è stato scavalcato ed ignorato e viene evocato, ministro Speranza, nei momenti in cui nel Parlamento dovete passare. Anche oggi, lei ha avuto parole assolutamente garbate

del Parlamento, mentre un decreto-legge deve essere comunque convertito. Vi è stata una situazione caotica inaccettabile e confusionaria, anche di alcuni enti e anche di alcune strutture sanitarie, che noi rispettiamo, perché non siamo tra coloro che minimizzano che negano i problemi e tutt'ora siamo attenti e preoccupati. Seguiamo le affermazioni della comunità scientifica, perché non possiamo dare per scontato nulla. Tuttavia, noi abbiamo assistito, in fase anche recente, all'INAIL che diceva che sull'autobus si stava a un metro al ristorante a due metri, allo stabilimento balneare a quattro metri e poi le Regioni hanno costretto il Governo a rivedere decisioni che erano cervellotiche: il pericolo, infatti, non è diverso sull'autobus o allo stabilimento balneare. E sto parlando di un paio di mesi fa. Quindi, confusione, arroganza e approssimazione, anche perché il problema è stato di una serie di abusi, come è stato già citato in questo dibattito e come riporta la risoluzione

ricordava che lei può intervenire con ordinanza in casi di emergenza. Perché, allora, spaventare turisti ed operatori economici con uno stato di emergenza fino al 31 dicembre, come avevate annunciato, invece che intervenire, come potete fare, in base a queste leggi, che il professor Cassese ha ricordato a tutti, in base alla decretazione? *(Applausi)*. si determinino situazioni pericolose. Avete tutti i poteri come Governo, e nessuno contesterebbe l'uso dei poteri che lei ha come Ministro della salute i poteri che il Governo ha di emettere decreti. Quanto ci vuole a riunire il Consiglio dei ministri se c'è una situazione di emergenza? Oramai siamo abituati a riunioni via video, via *web*, che vengono fatte a livelli planetari. I Consigli europei si sono svolti via Rete; noi, per fortuna, abbiamo mantenuto mantenuto l'abitudine del voto fisico in Aula. Tuttavia, non ci sono scusanti; c'è un'emergenza. Avete i poteri, gli strumenti e la tempistica per riunirvi nel giro di minuti e assumere decisioni. Quando Conte ha preso decisioni sbagliate ci ha messo pochi secondi a invadere le televisioni e stare ore e ore sforando gli orari dei telegiornali. *(Applausi)*. Siamo d'accordo che non si debba abbassare la guardia, crediamo che gli strumenti vadano usati in maniera appropriata. Oggi siamo qui a discutere di una proroga al 31 luglio; ci sarà, poi, l'occasione successiva in cui Presidente del Consiglio chiarisca in Parlamento: il 31 dicembre, il 31 ottobre, ma non è un negoziato politico; è una decisione che andrebbe assunta sulla base di evidenze scientifiche. Abbiamo grande rispetto per la comunità scientifica e per i virologi, però quando vediamo che Emiliano usa il suo virologo di fiducia come candidato alle elezioni, beh, ci chiediamo dove sta il trucco, dove sta lo scienziato e dove il candidato. *(Applausi)*. Siamo sottoposti a conflitti di competenze, conflitti di attribuzione, conflitti di potere. Dopodiché, il virologo va in televisione, poi si candida e non si capisce. Sarà uno? Non so gli altri; faremo il monocolore dei virologi, ripeto, pur rispettandoli. Non ripercorro qui la storia: mascherine che c'erano o che non c'erano, i congiunti, che non si capiva giuridicamente quale categoria del diritto fossero. Vi dirò di più: c'è un rischio di seconda ondata? conosciamo i Paesi, i luoghi dove oggi c'è il virus. E, allora, invece di attendere impotenti, si assumano decisioni verso quelle realtà, anche nelle sedi internazionali dove l'Italia deve far valere la sua voce. parte, se in qualche Paese c'è perfino il traffico dei certificati falsi che attestano l'immunità di una persona, interveniamo con quei Paesi. Non voglio nemmeno citarli, ma li avete letti. Volete estendere l'emergenza fino al 31 dicembre o al 31 ottobre e non andate in soccorso della Sicilia e della Calabria dove l'emergenza immigrazione sta dilagando. Facciamo nostro l'appello del presidente Santelli e del presidente Musumeci che hanno chiesto interventi adeguati. Sulle coste della Calabria e della Sicilia vogliamo le navi dei turisti, non le navi della quarantena per l'arrivo di clandestini in quantità, che già si annunciano. *(Applausi).* Oggi leggevamo sui giornali i soliti rapporti fondati dei Servizi di sicurezza che parlano della Libia, delle 20.000 o 30.000 persone pronte a sbarcare. Aspettiamo che la Calabria e la Sicilia, che hanno contenuto la pandemia, anche per la saggezza dei loro amministratori regionali, siano sommerse da questi problemi? Noi vorremmo sbarchi virtuosi di turisti, che non arrivano. Allora noi teniamo le porte aperte ai clandestini e teniamo le porte chiuse ai turisti. Andate a vedere a 50 metri da qui: hanno richiuso bar e ristoranti che avevano appena aperto perché c'è una crisi profonda. Volete la condivisione? Abbiamo dato voti decisivi per lo scostamento di bilancio, che è servito anche - lei le ha citate oggi, ministro Speranza - per le assunzioni della sanità: 29.000 - cito a mente - se ho sentito bene. è stato possibile anche per l'uso di quei fondi. I voti di tutto il centrodestra unito sono stati decisivi, ma non ci avete chiamato neanche un secondo a condividere le priorità su come utilizzare i soldi dello scostamento di bilancio.

probabilmente maggioritaria nel Paese, ed esigiamo rispetto quando si devono assumere le decisioni, non essere invitati dopo l'ultima giornata degli stati generali, dopo le archistar, i cantanti, dopo tutti quelli che, per carità, hanno diritto di dire la loro. Noi abbiamo un mandato per dire la nostra. Quindi abbiamo presentato una risoluzione perché siamo preoccupati per una seconda ondata e al Parlamento europeo proprio ieri l'onorevole Tajani e altri colleghi di Forza Italia hanno presentato un'interrogazione per richiamare l'Europa alle sue responsabilità sui controlli dei confini esterni d'Europa. Infatti, se in Libia abbiamo stanziato 110 milioni di euro europei per una serie di misure di supporto a quelle autorità, dobbiamo esigere il controllo delle coste della Libia, affinché non siano il luogo di partenza non sono di clandestini, ma a questo punto anche di pericoli sanitari.

gestiamo l'emergenza dove c'è e non annunciamo l'emergenza dove non c'è per creare un'immagine negativa e sbagliata del nostro Paese. *(Applausi)*. Avreste fatto meglio, colleghi della maggioranza e del Governo, ad accogliere la nostra risoluzione, che contiene considerazioni fondate e di buon senso. Non abbassiamo la guardia; non siamo qui a dire, come ha fatto Zingaretti in una giornata sfortunata, andate sui Navigli, mangiate e bevete. Siamo stati prudenti in tutta la fase di questa emergenza. Il presidente Berlusconi nei contatti internazionali con l'Unione europea ha sollecitato quegli strumenti - ma ne discuteremo un'altra volta - che servono. Mi auguro che le trattative sui fondi europei che Conte sta conducendo si concludano meglio di quanto oggi abbiamo letto sui giornali. Non mi è sembrato di grande successo il recente ma siamo preoccupati per la confusione che avete seminato. Siamo preoccupati per l'anno scolastico che riprenderà in maniera confusa. Poi, se uno critica il Ministro dell'istruzione è sessista. Noi non la riteniamo adeguata indipendentemente dalla sua collocazione politica o dal fatto se sia uomo o donna. Si potrà fare una critica, altrimenti siamo al sessismo alla rovescia, per cui uno non può criticare una persona. La ritiriamo inadeguata e lo sapete. Avete affiancato il Commissario avete preso delle misure; aspettiamo i banchi monouso, poi faremo i banchi monodose che butteremo il giorno dopo; non so che altro dovremmo attendere come invenzione. La scuola deve riaprire. *(Applausi)*. Concludo, Presidente: lo *smart working* deve essere una facoltà del progresso, non la desertificazione delle città, perché stanno morendo negozi, commercio, attività produttive. Allora, un conto è il progresso che ci consentirà l'uso di tecnologie, ma non è accettabile che l'Enel tenga a Roma la sede chiusa fino al 31 marzo. Lo sa, Ministro? *(Applausi)*. Quale emergenza ci sarà il 31 marzo? Avete la sfera di cristallo?

C'è un pericolo? Allora lo si programmi. Se il pericolo si è ridotto, riapriamo gli uffici e le città, perché oltre al pubblico impiego - che noi rispettiamo e stimiamo - c'è il commercio, i ristoranti e i pubblici esercizi, un'economia che deve vivere e che non può essere condannata a morte in tutte le città città italiane. Avreste fatto meglio ad ascoltarci. Il rispetto, ministro Speranza (lo dica anche al presidente Conte), non deve essere la circostanza del momento parlamentare; deve essere la pratica quotidiana della democrazia. Noi ci siamo, noi contiamo, noi vogliamo far valere il parere di milioni di italiani che rappresentiamo.

di parlare con serietà agli italiani. Devo dire che lei nei mesi di emergenza è stato uno dei Ministri presenti, puntuali, che rispondeva, mentre altri si sono eclissati. Quindi non c'è nessun pregiudizio politico, però non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi, sotto ricatto o sotto terrore per altri mesi in base al nulla. Ieri sono stati fatti 41.867 tamponi; i positivi sono stati solo 114. Nelle terapie intensive, per fortuna, sono rimaste solo 60 persone in tutta Italia. Fra i positivi, peraltro, 28 ce li hanno mandati in regalo con gli sbarchi in Sicilia e altri 11 con gli sbarchi in Calabria: almeno questi potreste fermarli? *(Applausi)*. Abbiamo problemi coi positivi italiani, almeno i positivi del resto del mondo possiamo evitarceli? Se c'è un Ministro dell'interno, che si faccia sentire, si faccia valere, si faccia vedere. *(Applausi)*. Il fatto che la situazione - grazie ai medici, al personale sanitario e agli italiani - sia sotto controllo non è dei sovranisti; non è di Salvini, di Orbán, di Trump, di Putin. Il pericolosissimo dottor Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha osato dire: «Stiamo dando al mondo l'idea di essere ancora in pieno dramma, che tutti i sacrifici non siano serviti a niente. Mentre è vero il contrario: il Covid è stata un'emergenza ospedaliera, che oggi, lo dicono i numeri, è finita». Smettetela di terrorizzare l'Italia e gli italiani. *(Applausi)*. Smettetela di vendere l'Italia al mondo come «il lazzaretto». Il virologo Massimo Clementi parla di una proroga come di un'incredibile forzatura; il primario di anestesia del San Raffaele, dottor Zangrillo, parla di una malattia uniformemente scomparsa dal contesto nazionale; il noto costituzionalista, leghista, salviniano e sovranista, Sabino Cassese definisce la proroga come inopportuna, perché il diritto eccezionale non può diventare la regola che le sue conseguenze negative per la società e per l'economia creano tensioni e bloccano l'economia. Rischiate di fare più danni per fame di quanti non ne abbia fatti il virus negli ospedali. *(Applausi)*. Per rispetto dei 35.000 morti, non potete tenere un Paese sotto ricatto. Il solo annuncio, la sola ipotesi di una proroga, sia essa al 31 dicembre o anche al 31 ottobre, senza nessun motivo scientifico, sta causando un danno di decine di miliardi di euro all'economia italiana. Chi paga? Chi risponde? Conte? Toninelli? Anche perché il dibattito surreale che si sta svolgendo sulle autostrade - su cui ancora oggi non pare che abbiate deciso nulla - vede, ancora oggi, non in una giornata di festa in cui la gente va in giro per il *week-end*, 13 chilometri di coda sulla A7 e 9 chilometri di coda sulla A9. Vi svegliate sbloccando le autostrade o no? Gli unici che stanno facendo un regalo ai Benetton sono coloro che stanno bloccando la Gronda di Genova che i Benetton dovrebbero pagare con 4 miliardi di euro. Voi state bloccando il Paese per i vostri pregiudizi. Gli unici che stanno facendo un regalo ad Autostrade per l'Italia sono al Governo. Ve lo chiediamo per cortesia: fate qualcosa. *(Applausi)*. In questi mesi, quante visite mediche sono saltate? Quante operazioni sono saltate? In questi giorni, quanti processi, non per grandi nomi, ma per semplici cittadini italiani, sono stati rinviati di anni? Va bene lo *smart working* e il lavoro da casa, ma spero che i magistrati tornino a lavorare sul posto di lavoro il prima possibile e a produrre. *(Applausi)*. A produrre sentenze, a produrre lavoro, a produrre giustizia. 6.000 farmacie sono a rischio di chiusura: 6.000 su 19.000, non solo in centro a Roma e Milano, ma nei paesi. Se in un piccolo Comune chiude una farmacia è un disastro, quindi vi preghiamo di ascoltare i farmacisti, di ascoltare noi e di fare qualcosa. Ci sono 10.000 medici laureati senza specializzazione; allo sforzo che avete fatto, se si aggiungono 4.000 borse in più, andiamo a eliminare il pregresso, ricordandoci, però, che da qui al 2025 andranno in pensione altri 30.000 medici. E non - come qualche fenomeno di giornalista ignorante ha scritto - per colpa di quota 100. Ricordo agli scettici di quota 100 che se non avessimo dato la possibilità di andare in pensione a 300.000 italiani, il virus avrebbe fatto anche altre vittime. E se qualcuno, fra i banchi del

Il modello Genova per velocizzare le opere pubbliche è contenuto in disegni di legge. A proposito di sanità, lei ha parlato di vaccino, che va bene. Io mi domando, però, perché si sia taciuto

Onore al dottor De Donno e a chi sta combattendo anche contro interessi economici che magari ci sono anche da queste parti. Quanto alla scuola,

Non è qua presente, ma lo è nello spirito e le faccio un appello. Ministro Azzolina, si dimetta, per cortesia: non è in grado di gestire la scuola italiana. La CISL denuncia 85.000 cattedre vuote. La proposta della Lega è di stabilizzare alcuni dei 200.000 precari che sono con i nostri figli da anni. Avete nominato il geniale commissario alle mascherine commissario alla scuola. Ma mi spiegate come uno che non ha portato le mascherine in Italia potrebbe riaprire le scuole dei nostri figli in sicurezza? *(Applausi)*. Non potete fargli fare qualcos'altro? Evidentemente, meno sono capaci, più sono promossi dal vostro punto di vista. I problemi sociali, di cui anche lei ha parlato, sono - ahimè

aggiornando i dati reali, i famosi 400 miliardi di euro che le banche avrebbero gentilmente donato agli imprenditori italiani sono fermi a 51. Il *bazooka* è un fucile ad acqua scarico. Se milioni di imprenditori, artigiani, partite IVA e commercianti sono andati in banca e tornati a casa con è perché il decreto sulle banche lo avete scritto con i piedi. Potete riscrivere il decreto liquidità aiutando i cittadini e non le banche? Altrimenti sarà un problema che ci ritroveremo nelle piazze. cento delle famiglie ha problemi con il mutuo, e sarà un problema sociale. C'è un abuso di psicofarmaci, e sarà un problema sociale. cento dei bimbi e minori ha problemi psicologici, e sarà un problema sociale. Nonostante questo, incredibilmente, avete confermato che lunedì 20 luglio

al lavoro pubblico da casa, a me fa piacere per i dipendenti pubblici che da qui al 31 dicembre potranno avere questa possibilità.

una riflessione che riguarda lei e tutti noi.Sono usciti i dati sui bambini che non nascono più: 420.000 nati l'anno scorso e nel 2021, se la politica non fa qualcosa e non si dà una svegliata, scenderemo sotto quota 400.000. È questo il dato sociale ed economico devastante per il nostro Paese, e non il 3 per cento *deficit*-PIL, lo *spread.* Se non nascono bambini - e l'Italia ormai è il secondo Paese più vecchio al mondo - è un problema. Mi auguro che nel decreto rilancio ci siano attenzione e sostegno economico anche per coloro che aiutano le mamme a diventare mamme e i papà a diventare papà.

alla - per loro nobile, per me indegna - battaglia per la legalizzazione delle droghe, dedichino altrettanta attenzione alla vita. Questo deve essere un Parlamento che si occupa di vita e non di droga e di morte. Smettetela di spaventare gli italiani, italiani, di tenerli chiusi in casa: gli italiani vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. Viva l'Italia, viva la vita e viva la libertà. Ministro, per favore, dia retta al Paese e non a qualche pseudo-virologo che ha suoi interessi privati o a qualche Ministro che non vuole perdere la poltrona. Grazie e buon lavoro.

prendo la parola in quest'Aula pensando a tutto ciò che è successo da fine febbraio ad oggi, perché qualcuno - sicuramente l'ultimo che ha parlato prima del sottoscritto - sembra averlo già completamente dimenticato. Voglio dire una cosa, Presidente: questo non è un Governo che si tira indietro. Non si è tirato indietro quando si è trattato di fare scelte dure, difficili, in quel periodo contestate anche da alcuni Paesi europei, come è stato il *lockdown*, mentre altri irresponsabilmente chiedevano di riaprire tutto. Non si è tirato indietro quando si è trattato di smentire menzogne - ahinoi quotidiane - come quella sul MES, che è uno strumento ratificato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2011, per mano di un Governo guidato da Silvio Berlusconi con dentro la Lega di di Salvini e Fratelli d'Italia. *(Applausi)*. Non si è tirato indietro nemmeno sulle scelte che si devono prendere sulla gestione delle nostre autostrade; ne ha parlato anche ora il *leader* della Lega e sappiamo benissimo - e io forse più di tutti che la Lega non è mai e poi mai stata d'accordo a revocare la concessione ad ASPI. A differenza delle menzogne quotidiane del *leader* di questo partito, non l'ultimo leghista arrivato, ma il Presidente della Commissione trasporti della Camera dei deputati, il leghista Morelli, lo ha dichiarato a chiare lettere pochi giorni fa in TV. TV. Siamo completamente stufi di queste menzogne. Ma veniamo a noi. Prorogare le misure già adottate per evitare la diffusione del coronavirus è sicuramente, signor Ministro e Governo, la scelta più giusta. Lo è per il MoVimento 5 Stelle. Lo sappiamo bene e lo sanno soprattutto i cittadini lombardi, come sono io stesso, che hanno sofferto più di tutti le devastanti conseguenze del coronavirus.

casi accertati di Covid. E chissà quanti altri ce ne sono stati e chissà quanti morti da Covid ci sono stati, ma non sono stati ovviamente sottoposti a tampone e non lo sappiamo. Sono decedute ad oggi 16.760 16.760 persone, su un totale in Italia di 34.984 persone che hanno perso la vita: una vera ecatombe.

toccato un *record* di 230.000 contagi in un solo giorno. Chi soffre, in particolare, ahinoi? Gli Stati Uniti e il Brasile soffrono, come abbiamo sofferto noi in Italia, ma con una piccola, grande differenza: lì

Come non ricordare che il presidente degli Stati Uniti Trump, nonostante il coronavirus avesse già contagiato oltre 3,3 milioni di persone e fatto 135.000 vittime circa, ha indossato per la prima volta la mascherina in pubblico due giorni fa. due giorni fa. In Brasile, da fine maggio, si registrano più di 1.000 morti al giorno, con un totale di oltre 72.000 decessi. È il secondo Paese solo dopo gli Stati Uniti;

tutti devono morire, nella più totale irresponsabilità *(Applausi)*. È l'esatto opposto di quello che è stato fatto in Italia grazie al presidente Conte e a questo Governo. questo è ciò che è accaduto in alcuni Paesi del mondo, ma non in Italia, dove, nonostante a febbraio ci fosse qualcuno che diceva che Milano doveva ripartire, questo Governo ha scelto invece la strada della responsabilità, adottando misure che ci hanno riconosciuto in tutto il mondo. Quando la Lega voleva riaprire tutto, c'è chi ha pensato a chiudere - e ci è voluto coraggio

come i bergamaschi non dimenticheranno mai i mezzi militari uscire dalla città carichi di feretri; i lombardi non dimenticheranno mai loro nonni

nemmeno oggi che i contagi sono diminuiti, ma non scomparsi. Non dobbiamo dimenticare che, se avesse governato chi a fine febbraio voleva tenere tutto aperto, avremmo i numeri degli Stati Uniti e del Brasile.

ancora una volta questo Governo perché sta scegliendo la strada della responsabilità onestamente spaventa, e parecchio, soprattutto quando queste critiche arrivano da parte di chi ha governato Regioni come la Lombardia dove i disastri commessi nella gestione della sanità da parte della politica sono sotto gli occhi di tutti.

Per non parlare ovviamente dei 37 miliardi di tagli circa operati in dieci anni al Servizio sanitario nazionale, che però abbiamo cancellato - è vero - da quando il MoVimento 5 Stelle sta al Governo, invertendo la rotta e tornando a investire nella sanità pubblica, come confermano i nuovi stanziamenti inseriti nei decreti cura Italia e rilancio. Abbiamo raddoppiato i posti letto in terapia intensiva e aumentato quelli in subintensiva. Abbiamo previsto più assunzioni e rafforzato l'assistenza domiciliare. *(Applausi).*

anche se una cura non c'è ancora: non abbiamo ancora un vaccino e, quindi, l'allerta deve rimanere massima e immediate devono essere le misure che dovremo mettere in campo laddove ce ne dovesse essere estrema necessità. Ed ecco giustificato il sì del MoVimento 5 Stelle alla proroga dello stato di emergenza. Certo, sappiamo benissimo che dopo la crisi sanitaria è scoppiata una crisi economica; lo sappiamo perché siamo intervenuti. Questo Governo non ha perso tempo nemmeno lì: cassa integrazione, *bonus* per le partite IVA, *bonus baby-sitter*, reddito di emergenza *(Applausi)* per chi per l'emergenza ha perso tutto e fondi ai Comuni per aiutare chi è rimasto in ginocchio. Sono stati stanziati 80 miliardi. Avete idea di quante risorse siano? Parliamo di uno sforzo economico superiore a due leggi di bilancio e lo abbiamo fatto, sì, nel modo migliore in cui era possibile farlo. Certo, non potevamo cambiare la burocrazia italiana con una bacchetta magica, ma lo stiamo facendo adesso con il decreto semplificazione. Poi siamo andati in Europa grazie al lavoro certosino del presidente Conte, oggi si parla di *recovery fund*, cioè si parla di oltre 170 miliardi che arriveranno all'Italia. E a chi fa polemica anche su questo, a chi fa polemica anche sui 170 miliardi che arriveranno all'Italia, all'Italia, facciamo un semplice appello: basta, basta, basta polemiche e propaganda; almeno su questo si dovrebbe smettere di fare la guerra a questo Governo e con senso di responsabilità dare una mano all'Italia e agli italiani a vincere

macchina del fango? Vediamo niente poco di meno che l'alleato di Salvini in Europa, Geert Vilders, sollevare un cartello con sopra scritto: «Non un centesimo all'Italia». Begli alleati! Chissà che rivoluzione a favore degli italiani avrebbero fatto se fossero stati al posto di Conte. Vi direi: oltre al danno la beffa; ma c'è solo la beffa, perché fortunatamente Salvini al Governo non ci sta e il danno l'abbiamo evitato. Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle ha a cuore i lavoratori, le imprese, le famiglie, così come abbiamo a cuore la salute dei cittadini. E per questo votiamo sì alla proposta di risoluzione che proroga le misure di contenimento del virus, perché evitare il contagio da coronavirus deve rimanere la nostra priorità. Qui si tratta non di limitare la libertà di nessuno - come ha detto poco fa chi mi ha preceduto - ma di incentivare quelle misure, come lo *smart working*, che si sono rivelate fondamentali nei mesi di emergenza. Prevenire è l'arma più forte che abbiamo, mentre sfruttare le preoccupazioni dei cittadini, facendo credere falsamente che li vogliamo rinchiudere nuovamente in casa - è falsa questa affermazione di poco fa - è un atto vile

mesi. Però mettiamo dei puntini sulle i. A noi del MoVimento 5 Stelle la propaganda non interessa *(Commenti)*. A noi le menzogne non interessano.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

recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»,

In relazione a quanto riferito dal senatore Pesco, l'esame del disegno di legge è rinviato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

La Provincia di Nuoro nasce nel 1927. Nuoro è una città ricca di musei, tra cui quello dedicato al premio Nobel Grazia Deledda, circondata da una natura di inenarrabile bellezza e da numerosi siti della civiltà nuragica. Tuttavia, ha il triste primato di non avere una linea ferroviaria statale. Alla città di Nuoro e all'intera Provincia è negato un dignitoso servizio pubblico essenziale su rotaia, essendo le stesse dotate unicamente di una linea a scartamento ridotto risalente ben al 1889, oggi di proprietà dell'Azienda

Soltanto qualche anno fa un treno all'apparenza moderno è stato sostituito alle vecchie littorine ma, poiché le rotaie sono rimaste le stesse, questo viaggia lentissimo. Occorre che l'azienda Rete ferroviaria italiana (RFI) preveda una nuova linea ferroviaria che sostituisca il tratto a scartamento ridotto e colleghi Nuoro al porto e all'aeroporto di Olbia, favorendo la libera circolazione delle persone e delle merci e, quindi, anche i flussi turistici nelle zone interne della Sardegna. La riconversione della linea Nuoro-Macomer e la nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia rappresenterebbero dunque l'indispensabile soluzione per porre un argine all'isolamento e allo spopolamento dei paesi della Provincia di Nuoro, diventati una vera e propria isola nell'isola. Si apprende dal contratto di programma con RFI per gli anni 2017-2022 che l'ipotesi di una tratta ferroviaria nuova che unisca la città di Nuoro alla città di Olbia

la presenza della strada statale 131 non dovrebbe influire in alcun modo sulla previsione di una nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia, in quanto i benefici oggi sono da valutarsi in termini di utilità sociale e di sviluppo turistico. La logica costi-benefici, se intesa solo

che conta una popolazione limitata numericamente, ma disseminata in un territorio isolato e vasto e che pertanto necessita di collegamenti efficienti, con porto e aeroporto, presenti invece a Olbia, per potersi sviluppare economicamente, soprattutto nelle zone interne. Concludo, signor Presidente, auspicando un intervento immediato sia della Giunta regionale sarda, per quanto riguarda la cessione da parte di ARST della tratta ferroviaria Nuoro-Macomer a RFI, sia del Governo che ponga fine all'isolamento di Nuoro e della sua Provincia, garantendo una nuova linea ferroviaria statale

Presidente, onorevoli colleghi, oggi porto all'attenzione di quest'Assemblea l'ultima inchiesta in ordine di tempo che vede coinvolto il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), ente concessionario dal novembre 2000 delle tratte autostradali A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania e della Siracusa-Gela ancora in costruzione, facente parte dell'asse viario europeo E45. L'indagine in questione, coordinata dalla procura della Repubblica di Messina, è stata chiamata «Fuori dal tunnel» e mai denominazione fu più azzeccata. È notizia di pochi giorni fa, infatti, quella dell'arresto di funzionari del consorzio e di alcuni imprenditori per corruzione,

appalti truccati che riguardano lavori effettuati negli ultimi anni lungo il tratto autostradale di competenza del CAS (A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania) e irregolarità che sarebbero emerse anche nei lavori eseguiti per la riapertura della galleria di Sant'Alessio sull'autostrada A18 Messina-Catania. La procura, in particolare, avrebbe ipotizzato la sussistenza di gravi anomalie nella realizzazione di questi interventi, con particolare riferimento anche a un importante sistema di sicurezza delle gallerie. A seguito di questa indagine, l'ennesima, che riguarda il CAS, ho predisposto un'interrogazione rivolta al ministro delle infrastrutture

e sull'adeguatezza di questo ente, in un'ottica di revisione della concessione, anche a livello nazionale. Reputo che sia arrivato il momento di valutare l'immediato ritiro della concessione,

come, dal 2014 al 2017, siano stati affidati ben 220 incarichi a un solo legale di Messina e 71 a un avvocato di Palermo: una ulteriore, preoccupante conferma della mancanza di trasparenza anche negli affidamenti delle consulenze da parte dell'ente che ha un contenzioso per oltre 200 milioni di euro. Vorrei porre all'attenzione dell'Aula una ulteriore indagine degli ultimi giorni che riguarda proprio il tratto autostradale Messina-Palermo, tra i comuni di Milazzo e Rometta. Sono state sequestrate due strutture che erano a rischio crollo. per l'omessa vigilanza e la mancata manutenzione di quei viadotti la procura della Repubblica ha iscritto ulteriormente nel registro degli indagati alcuni tecnici del CAS e l'attuale direttore generale. «Fuori dal tunnel», quindi, è l'ultima di una serie di indagini che hanno colpito questo ente ad altissimo tasso di corruzione e che presenta fortissime carenza a livello strutturale e organizzativo. Il CAS è, a questo punto, l'emblema dello spreco di denaro pubblico compiuto sulla pelle e sulla sicurezza dei siciliani. Per questo chiediamo di uscire fuori dal tunnel, il tunnel dell'illegalità.

una preghiera laica a lei, signor Presidente. La interrogai già cinque mesi fa, quando venne arrestato Patrick Zaki in Egitto per aver pubblicato dei *post* e aver espresso le sue idee, nonostante fosse in Italia, a Bologna. Oggi la sua detenzione illecita è stata prorogata di altri quarantacinque giorni. Zaki è stato spostato nella prigione di Tora, dove Amnesty International ha ha dichiarato che è morto da poco un giornalista detenuto per Covid. Vorrei sapere quanto altro dobbiamo consentire agli egiziani di fare sulla pelle di quel ragazzo nell'assoluto mutismo di quest'Aula e di tutte le altre aule istituzionali. Alcune si sono pronunciate: il Comune di Milano ha dato a Zaki la cittadinanza onoraria, a Zaki la cittadinanza onoraria, così come Bologna e Napoli. Io, signor Presidente, le avevo chiesto di autorizzare una missione e lei mi ha risposto, correttamente, che non avrebbe potuto farlo. Io ho interloquito, su suo consiglio, con il Presidente della Commissione esteri e con il Presidente della Commissione diritti umani. Mi è stato promesso che il nostro ambasciatore si sarebbe fatto carico del problema. Oggi Zaki è stato spostato in un carcere dove rischia di morire. Io le chiedo, e la prego, lei che difende giustamente le prerogative di quest'Aula davanti anche delle possibili distrazioni del Governo, di interrogare il Ministro degli esteri su questo. Non mi spingo a perorare ciò che chiede la famiglia di Giulio Regeni, che dice che dovremmo nuovamente ritirare l'ambasciatore, ma il nostro ambasciatore si faccia sentire per la vita di questo ragazzo e perché quest'Aula abbia una spiegazione sul perché continuiamo a interloquire con l'Egitto nonostante le continue violazioni dei diritti umani.

Quindi, quando le ho dato una risposta, è proprio perché li avevo fatti. Comunque, proverò a ripeterli. Le assicuro, però,

stimato collega condannato al consiglio disciplinare per una vicenda che ha scosso tutto il settore medico. Il professor Mario Di Fiorino, primario di psichiatria presso l'ospedale Versilia, Regione Toscana, ha espresso, via *social*, commenti e preoccupazioni circa l'organizzazione dei laboratori sul territorio per assolvere con tempestività le analisi dei tamponi e, soprattutto, la necessità che tale organizzazione garantisse un intervento adeguato in caso di positività

alla psichiatria, della quale il professor Di Fiorino è responsabile. Signor Presidente, stiamo parlando di realtà che hanno rappresentato, fino ad oggi, il più alto rischio di diffusione di contagio del virus tra pazienti e personale sanitario. Mentre l'OMS e il Ministro della salute annunciavano l'allarme pandemia, per assurdo, la direzione aziendale ASL-Toscana Nord Ovest ha ritenuto che: ritenuto che: «il pensiero espresso dal professore possa creare, nella popolazione già provata in un momento di emergenza sanitaria, un senso di tristezza, incertezza e sfiducia nei confronti del Servizio sanitario pubblico». Colleghi, il pensiero! È per questo che che l'ASL Toscana è intervenuta con differimento del professore al consiglio disciplinare. In sostanza, il collega Mario Di Fiorino, psichiatra, è stato deferito al consiglio di disciplina perché, in piena pandemia, aveva richiesto richiesto che l'ospedale fosse messo nelle condizioni di poter eseguire i tamponi. Ma pensavano forse di guarire i pazienti con omeopatia o fiori di Bach? Anche questa volta, il Sistema sanitario della Regione Toscana non si è smentito. Nella gravità del momento, ha voluto colpire senza pietà il servizio medico psichiatrico. Io sospetto che, se l'appello fosse giunto da un qualsiasi virologo, immunologo, infettivologo o epidemiologo, "ultimominutologo" da prima serata TV, anziché da parte del servizio psichiatrico, la risposta avrebbe avuto altre attenzioni: un peso, due misure. Eppure, la questione sollevata dal professor Di Fiorino, contrariamente a quanto riportato dall'azienda sanitaria, dimostra invece una particolare sensibilità alle problematiche concrete relative alla struttura sanitaria, soprattutto dei pazienti e degli operatori psichiatrici, che, nonostante la martellante cronaca che tutti i giorni abbiamo la disgrazia di ascoltare, continuano a essere anime senza voce. Per questo, io non smetterò di appellarmi, anche in questa sede, per il loro umano diritto alla cura e non solo per il Covid-19.